il disegno di legge n. 1048 reca la delega al Governo per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. L'atto è stato approvato in prima lettura alla Camera il 27 febbraio 2024 e trasmesso il successivo 28 febbraio al Senato. L'articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di florovivaismo nei termini appena esposti. L'adozione dei relativi decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. L'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Più in particolare, le lettere dalla *a)* alla *v)* del comma 1 indicano al Governo la necessità di disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica; definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l'articolo 2135 del codice civile e con le disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 2004, prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo di livello dirigenziale, non generale, presso il MASAF; prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali; elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico che individui specifiche azioni di intervento; predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; pianificare e istituire a livello nazionale piattaforme logistiche per macroaree; prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli destinati al florovivaismo in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica, nonché della loro sostenibilità ambientale; effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto dei livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo a cura del MASAF l'istituzione di un marchio unico distintivo; qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo; definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento; prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori; definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche; disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato; definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale quali elementi di promozione delle attività di forestazione, soprattutto nei confronti dei Comuni di minori dimensioni; prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica. L'articolo 3 indica il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che gli schemi predisposti dal Governo ai fini dell'esercizio della delega siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un ufficio per la filiera di florovivaismo presso il MASAF e stabilisce che le ulteriori disposizioni delegate non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. Per un approfondimento delle disposizioni appena sintetizzate si fa rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici e disponibili in Aula in formato cartaceo e sul sito Internet dell'Amministrazione. Vorrei aggiungere inoltre una breve considerazione, ritenendo il tema dei provvedimenti in esame importantissimo per i protagonisti del settore. Il florovivaismo, infatti, è un settore che attendeva da tempo che attendeva da tempo una legge volta a sostenere e promuovere la produzione. Era necessario un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Ed è proprio il compito che questa legge delega assegna al Governo. La produzione florovivaistica italiana è uno dei settori più importanti del nostro *export* e, di conseguenza, uno di quei settori che favorisce i dati positivi della nostra economia. L'Italia è la seconda esportatrice europea del prodotto orto-florovivaistico, dietro ai Paesi Bassi e davanti alla Germania ed alla Spagna, e vale 1,23 miliardi di euro come valore di produzione. In ogni Paese europeo e nei principali Paesi extraeuropei, la floricoltura italiana ha saputo imporsi per l'alta qualità e la tipicità delle produzioni di piante e di fiori. Sebbene l'andamento in termini economici abbia faticato a crescere negli scorsi anni, riuscendo ad affermarsi però nel biennio 2021-2022, il valore della produzione delle aziende florovivaistiche italiane rappresenta oltre il 5 per cento del valore della produzione agricola totale e deriva, per il 50 per cento, dal comparto di fiori e piante in vaso, mentre il restante 50 per cento da piante, alberi e arbusti destinati al vivaismo. In Europa, l'Italia è tra i primi Paesi per dimensione della superficie destinata al vivaismo e alla coltivazione di piante e fiori in genere. Il favorevole clima italiano e la selezione di specie particolarmente resistenti alle alte temperature estive, nonché alla carenza di acqua, come quelle tipiche della flora mediterranea, sono le basi del riconoscimento e del concetto di qualità che che contraddistingue la produzione italiana delle piante da esterno: quindi, non solo delle belle piante, ma anche e soprattutto adatte ad un giardinaggio sostenibile e più naturale. Il tutto, al passo coi tempi e con le più attuali linee di progettazione paesaggistica. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Licheri. Signor Presidente, saluto il Sottosegretario, i membri del Governo, le colleghe e i colleghi presenti. Devo dire, con dispiacere e con rammarico, che rileviamo che ci troviamo a discutere, ancora una volta, un provvedimento delega al Governo, soprattutto per un tema sul quale, come accade spesso, anzi sempre, il MoVimento 5 Stelle cerca di fornire un aiuto concreto con proposte emendative puntuali e precise, che però non sono state degnate di attenzione. Infatti, nessun emendamento dei 43 che abbiamo presentato è stato accolto: quindi, l'ennesimo schiaffo alla nostra attività parlamentare, alla funzione legislativa che continua, in maniera insistente, ad essere mortificata. Condivido con voi alcuni dati di questo settore perché, nonostante la mortificazione della nostra attività emendativa, crediamo che il settore crediamo che il settore continui a meritare, nonostante quello che abbiamo subito, la nostra attenzione. Non smetteremo assolutamente di farlo, farlo, perché il settore florovivaistico rappresenta per l'economia italiana e il *made in Italy* uno dei comparti tra più importanti, con il 5 per cento della produzione agricola totale e con una crescita dell'11,4 per cento. È un valore che ha superato, nel 2022, i 3,1 miliardi di euro. L'Italia, con questi risultati, è tra i primi

sotto il profilo sociale, architettonico e di tutela della biodiversità, soprattutto nei contesti altamente antropizzati. Tutti, quindi, riconosciamo l'enorme valore di questo settore, non soltanto sotto l'aspetto economico; ne riconosciamo le enormi potenzialità per la salute e per la transizione ecologica. Come dicevo, però, questo settore non è estraneo a una serie di criticità e di problemi. Gli operatori del settore devono confrontarsi infatti ogni giorno con l'aumento dei costi di produzione. Parliamo di fertilizzanti, imballaggi, gasolio per il riscaldamento delle serre e trasporto che si aggira intorno ad un più 28 e che ricade poi sull'aumento dei prezzi di vendita: in media, un più 11,3 per cento. Gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, quali la siccità e le alluvioni, distruggono intere produzioni. è poi l'aumento delle importazioni, ma soprattutto l'assenza di un piano nazionale che possa fare una certificazione e tracciare una rilevazione dei dati del settore. dunque, affrontiamo tutti questi problemi con una delega al Governo, l'ennesima iniziativa che definisce una cornice, un insieme di linee di intervento, ma che continua a lasciare molti spazi bianchi in questa pagina, con inevitabili ritardi. questo ricorrere a presentare una scatola vuota è un metodo che sta piacendo molto all'Esecutivo (è successo recentemente con l'autonomia differenziata): si traccia un perimetro e poi gli altri se ne devono occupare, gli altri devono riempire questa scatola. È un chiaro annuncio, una bandierina, l'ennesima bandierina che viene posta in questo caso su un settore che grida aiuto. Mi perdoneranno i colleghi campani, ma a Napoli c'è un modo di dire molto efficace: *facimm' ammuina*, cioè facciamo chiasso, creiamo disordine, ma poi i problemi restano. Nel testo si parla di strategia nazionale, ma è solo la somma di una serie di indicazioni generiche. generiche. Continua a mancare una visione, una direzione che ci dica cosa fare di interi settori della nostra economia, in questo caso del caro florovivaismo, che - è proprio il caso di dirlo - è un fiore all'occhiello del nostro Paese all'estero. Rispondiamo a queste richieste di aiuto con un piano d'intenti. non ci sono tante risorse, ma questo è un disco rotto, una colonna sonora che accompagna tantissime grandi idee di questo Esecutivo, anche se qualche risorsa è stata individuata e devo dire che il ministro Lollobrigida - lo dico con ammirazione - riesce sempre a trovare qualche soldino, se pensiamo a *staff* stellari e uffici. In questo caso il provvedimento prevede la nascita di un ufficio per la filiera del florovivaismo, Il florovivaismo ha subito enormi mutamenti negli ultimi vent'anni per stare al passo con le continue nuove esigenze di questo mercato e, proprio in virtù di tutti questi sacrifici fatti, gli addetti e le imprese del settore meritano un atteggiamento e provvedimenti responsabili che vadano dritti al cuore dei problemi. Tempo fa i colleghi della Lega avevano chiesto la procedura d'urgenza per rispondere

Se vogliamo valorizzare il patrimonio florovivaistico, così importante per il nostro Paese, dobbiamo lavorare per sostenere le imprese facilitando l'accesso al credito, monitorare, tracciare, semplificare tutte le procedure, salvaguardare salvaguardare il comparto dalla concorrenza sleale di altri Paesi, rinnovare gli impianti serricoli dismettendo quelli troppo vecchi, monitorare i prezzi, puntare sui territori, sulle specificità di ognuno di essi per esaltare le produzioni locali; spingere sulle intese di filiera per tutelare addetti e imprese; puntare sul valore sociale del florovivaismo, con particolare attenzione all'inclusione di soggetti fragili, e soprattutto stabilire i criteri di premialità per le aziende che hanno requisiti etici e di onorabilità. I fatti delle ultime ore, che hanno portato alla morte Satnam Singh, ma non solo, rendono ancora più urgente che i comparti dell'agricoltura e del florovivaismo rispettino criteri etici forti. I temi e le soluzioni ci sono, ma serve un atteggiamento serio, una volontà politica e non soltanto annunci. L'impegno deve essere di tutti, nessuno escluso. Noi non ci siamo sottratti a questo impegno; ripeto che la nostra attività emendativa è stata puntuale e precisa, ha cercato di rispondere alle esigenze del settore. Qui in Senato non abbiamo avuto la possibilità di procedere con le audizioni, ma questo non ci ha fermato. Abbiamo comunque ascoltato i rappresentanti della categoria e con i nostri emendamenti abbiamo cercato di riempire quei vuoti che, a nostro avviso, la vostra proposta continua a mantenere. La vostra proposta rimane, dunque, tale: una bella cornice; sicuramente la confezione è molto accattivante e affascinante, però per noi rimane una scatola vuota e aspettiamo di vederla riempita.

rispondo alla collega Licheri, che citava un vecchio adagio napoletano, *facimm' ammuina*, dicendo che l'obiettivo di questo provvedimento è proprio l'opposto: andare a regolamentare un settore e un comparto che è molto importante e che aveva bisogno di una normativa in tal senso. senso. È importante perché è una filiera trainante del *made in Italy* ad alta densità di investimenti e specializzazione, che da anni insegue un riconoscimento. È l'*identikit* del comparto florovivaistico, la cui produzione, come diceva anche prima la collega, nel 2022

La bilancia commerciale evidenzia anche un'annata positiva, con un 1,2 miliardi di vendite oltreconfine contro 890 milioni di *import* ed oggi, grazie a questo Esecutivo, il riconoscimento inseguito finalmente arriva. Il comparto del florovivaismo, infatti, con i suoi prodotti, rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo ed è ambito di forte presenza occupazionale e di competenza. Il settore, peraltro, è uno dei maggiori in ambito agricolo ad alta densità di tecnologia e di ricerca. Parliamo di un comparto dall'occupazione complessiva, compreso l'indotto, di oltre 200.000 persone. uno dei settori di punta del *made in Italy*, ma vive un momento difficile a causa di importazioni selvagge basate su concorrenza sleale e delle impennate dei costi di produzione. Questo provvedimento, con tutto quello che va ad inquadrare e regolamentare, serve anche a tutelarci dalla concorrenza sleale, facendo in modo che piante e fiori in vendita in Italia e in Europa rispettino le stesse regole su ambiente, salute e diritti dei lavoratori. I prodotti del florovivaismo sono utilizzati anche all'interno delle nostre città, contribuiscono al mantenimento dell'ambiente e al decoro delle aree verdi urbane e migliorano l'equilibrio ecologico all'interno dei nostri territori. I vari studi di mercato evidenziano che l'Italia è la seconda esportatrice europea del prodotto ortoflorovivaistico, dietro solo ai Paesi Bassi e prima di Germania e di Spagna. L'*export* tricolore ha raggiunto una quota di 1,23 milioni di euro come valore della produzione, anche questo dato in crescita sul 2021, sulla base di elaborazioni Istat ed Eurostat. A questo si ricollega anche un'impronta identitaria forte. Infatti il florovivaismo è tra le filiere di punta, come dicevo, del *made in Italy*, ovvero tra quei prodotti a saldo stabilmente positivo che notoriamente richiamano il nostro Paese dal punto di vista dell'immagine e che, con un valore di 980 milioni Grazie a tutto comparto, che negli anni delle limitazioni imposte dal Covid è stato messo in ginocchio. Il settore, infatti, ha dovuto affrontare numerose criticità, a partire dall'azzeramento della domanda da parte degli operatori del turismo e della ristorazione. gli operatori del settore, questa legge delega definisce l'architrave che rappresenta a sua volta una svolta, poiché chiarisce ruoli, competenze, forme giuridiche, interlocutori istituzionali e programmazione a partire da una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica, in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dall'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore. legge prevede, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura di un ufficio per la filiera che garantisca una gestione efficace del settore, la valorizzazione dell'attività e la predisposizione di un piano nazionale del settore. Per la prima volta, inoltre, si parla anche di filiere produttive di livello regionale. La premialità per le aziende florovivaistiche entrerebbe per la prima volta nei piani di sviluppo regionale, che hanno sempre visto il florovivaismo svantaggiato rispetto ad altri settori, comparto che si caratterizza anche per un forte potenziale ambientale e paesaggistico su cui la riforma intende puntare, riconvertendo gli impianti serricoli destinati a florovivaismo in siti agroenergetici. Per anni abbiamo subito le politiche avviate da Bruxelles, una rivoluzione ambientale che ha mostrato - e continua a farlo ogni giorno - tutte le sue incongruenze e tutte le sue follie. Tra queste c'è anche il fatto che proprio uno dei comparti che più possono dare un contributo in termini di riduzione delle emissioni e in vista degli obiettivi di neutralità climatica sia stato lasciato ai margini. E così, mentre tutti parlano, tacciano questo Governo di negazionismo, si riempiono la bocca di ambiente ed osannano l'Europa dei burocrati, chiedendone sempre di più anche nei simboli partito, noi realizziamo i fatti e lo facciamo a tutela dell'Italia, di chi lavora, di chi produce in maniera sana e non ideologica, per e con l'ambiente. Mi viene in mente quando, un paio d'anni fa, la von der Leyen proposte di piantare in Europa tre miliardi di alberi

prospettive senza coinvolgere i veri addetti ai lavori, quelli che noi oggi chiamiamo in causa per programmare la produzione vivaistica e per fare formazione e manutenzione. Quello del florovivaismo è un settore con 24.000 aziende in Italia. Può svolgere un ruolo di primo piano non solo sul fronte della forestazione, ma anche su altri decisivi ambiti contemplati nel PNRR, come i parchi agrisolari, l'agrivoltaico, le comunità energetiche, il teleriscaldamento da biomasse e così via; eppure prima di noi non è stato tutelato né chiamato in causa dai vari ambientalisti d'assalto. Siamo reduci da un'ideologia *green* che ha sfoggiato tutte le sue posizioni deliranti, anche nel Governo precedente a questo. Penso alle tante persone che hanno definito l'essere umano biologicamente un parassita, perché consuma energia senza produrre nulla, in un mondo progettato per 3 miliardi di persone. Ma nessuno mai ha chiarito la fonte di queste rivelazioni e cosa pensa di fare con i circa cinque miliardi di parassiti in eccesso. Vede, Presidente, bene l'ecologia, certamente, purché sia un'autentica ecologia umana, che rispetti innanzitutto la natura dell'uomo e, conseguentemente, anche tutto il resto del creato. Con questa legge delega noi facciamo esattamente questo, per tutelare prima di tutto chi lavora in questo comparto. L'uomo, nell'ambito biologico e dell'ambiente, noi non lo definiamo un parassita, mai, anzi lo difendiamo e lo facciamo lavorare.

Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti gli onorevoli senatori che hanno contribuito a portare in Aula oggi questo provvedimento importante. Non aggiungo altro a quello che è già stato detto da chi mi ha preceduto. Ci tengo a ringraziare - come dicevo - tutti gli onorevoli senatori, in particolare i membri della Commissione agricoltura, la relatrice e il Presidente. Ma soprattutto ci tengo a ringraziare pubblicamente tutti i nostri imprenditori e tutte le nostre aziende, che, nonostante in questi decenni non abbiano mai avuto una strategia nazionale su cui potersi appoggiare, hanno fatto di questo settore uno dei settori di eccellenza dell'agricoltura italiana, come anche i numeri indicati da coloro che mi hanno preceduto testimoniano.

i nostri uffici stanno già lavorando a una bozza, in modo da poterla condividere con tutte le associazioni del settore, perché è nostro interesse e nostro intento, anche per l'attenzione che vogliamo dare a questo settore, riuscire a stringere il più possibile i tempi per giungere finalmente a definire una strategia concreta e un piano di settore per il florovivaismo. Mi fermo qui perché non ho altro da aggiungere, ringraziando ancora tutti per il grande lavoro fatto.

un inserimento importante nel florovivaismo. Ben venga che nel disegno di legge sia previsto un intervento per individuarle e pianificarle, però vorremmo uscire

colpito duramente dalla crisi energetica di quel momento. Sappiamo benissimo che è un settore fortemente energivoro. Peraltro, si trattava di risorse anche eccessive rispetto alle esigenze delle 8.000 aziende che ne chiedevano l'attuazione immediata, tanto che quelle risorse poi sono state utilizzate anche per altro, perché oggettivamente erano sovradimensionate, ma in quella fase era giusto dare un sostegno al settore. Quindi non rappresenta del tutto la realtà dire che non c'è mai stato un sostegno a favore del florovivaismo, settore fondamentale per l'agricoltura. Il

al settore agricolo non ci fossero mai divisioni politiche o tentativi di dividere, perché credo che sia fondamentale che il sistema Paese, come ha fatto tante volte, si dimostri vicino agli interessi degli agricoltori, che sono il vero traino economico e il motore del Paese.

trova il sottoscritto, ma anche da sempre la Commissione, assolutamente favorevoli; non può che essere così, proprio nell'interesse superiore degli agricoltori e nell'interesse nazionale, in un settore

Chiedo ai colleghi che intendono lasciare l'Aula di farlo in silenzio per permettere alla senatrice Musolino di parlare. MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la legge delega che ci accingiamo a votare ha un percorso abbastanza lungo, viene da lontano e finalmente arriva alla sua definizione in Parlamento. È una legge delega con la quale sostanzialmente

riguardante il florovivaismo. È una legge ambiziosa, della quale sicuramente c'era necessità, proprio per dare ordine e sistema a un settore produttivo produttivo tra i più importanti per l'Italia, non soltanto in termini numerici, quantitativi e di volume dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la storia, la tradizione e il valore delle nostre capacità, apprezzate in tutto il mondo.

la volontà di realizzare un quadro normativo, in cui si tenga conto anche della tradizione e si cerchi di sviluppare e implementare questa tecnica e, conseguentemente, la produzione, è sicuramente apprezzabile ed è uno dei motivi per i quali posso anticipare fin da adesso Italia Viva-Il Centro-Renew Europe esprimerà un voto favorevole su questo disegno di legge. Ci sono anche altri aspetti che mi piace citare, perché contribuiscono a motivare questo voto favorevole.

rileviamo anche attraverso statistiche, non capiamo quali coltivazioni vanno meglio di altre, di cosa c'è più necessità e in quale

unico, di durata quinquennale, è sicuramente uno strumento apprezzabile, di cui vi era necessità. Allo stesso modo, è apprezzabile che finalmente si parli anche di filiere produttive dal punto di vista regionale, perché sono strumenti - anche questi - di programmazione, sviluppo e promozione che, all'interno di un piano nazionale, contribuiscono finalmente a dare organicità non soltanto dal punto di vista normativo, ma anche produttivo. In questo senso, anche la previsione dell'individuazione delle piattaforme logistiche (cioè pianificare e istituire a livello nazionale piattaforme logistiche per macroaree) è sicuramente un punto importante contenuto in questo disegno di legge.

il bene è nemico dell'ottimo, come dice talvolta il nostro Presidente del Senato, pertanto mi rammarico, ma questo non è un motivo sufficiente per esprimere un voto contrario. Invece, approviamo e siamo sicuramente favorevoli al fatto che venga finalmente data attenzione alle piattaforme logistiche, che è un punto fondamentale, soprattutto al Sud, grande produttore del florovivaismo, perché la mancanza di infrastrutture logistiche penalizza la produzione italiana. Poi diventa difficile trasportare le merci, esportarle o comunque farle viaggiare sul territorio nazionale. La piattaforma logistica è sicuramente un'apertura importante e uno strumento da non sottovalutare. Per questo

è probabilmente arrivata attraverso palme di importazione. Un marchio unico distintivo serve allora a fare una distinzione fra chi rispetta i criteri e chi non li rispetta e aiuta anche il consumatore a rivolgersi a chi effettivamente, rispettando le regole, magari deve spendere di più per garantire una produzione di qualità. Tuttavia, a quel punto il consumatore sa che, investendo su chi rispetta le regole, è garantito non soltanto nell'acquistare un prodotto di buon livello, ma anche nel fatto che i lavoratori che hanno realizzato quella produzione non sono stati sfruttati. E di questi tempi, proprio con le vicende che si sono verificate in queste ultime ore e di cui parleremo durante il *question time* sul caporalato, direi che questo è proprio importante e fondamentale. Occorre però che il marchio unico distintivo non sia soltanto

si faccia soltanto un uso strumentale, che non garantisce veramente il rispetto delle regole. Ben venga, a questo punto, la definizione delle figure professionali che operano nel settore del florovivaismo,

che possono contribuire non soltanto a formare una classe di operatori specializzati che aiuti gli imprenditori nelle coltivazioni, ma anche a sviluppare una cultura e una conoscenza del florovivaismo che è fondamentale recuperare

dell'energia elettrica, mentre questa tipologia di impianti darà un grande impulso anche all'agricoltura. Penso anche e soprattutto ai territori del Sud, dove la conversione degli impianti è fondamentale e dove vanno aiutati gli imprenditori che riescono a fare questa scommessa, perché ci credono e chiedono di essere aiutati. In questo senso anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fare contratti di locazione con agevolazioni commerciali per gli imprenditori agricoli per l'allocazione dei tanti terreni. Anche su questo, penso che tale tipo di delega debba anche incontrare altri provvedimenti e che debba anche intrecciarsi, per esempio, con il catasto terreni, perché ci sono tanti terreni abbandonati, che i Comuni non possono utilizzare, perché neanche li conoscono e non ne hanno neanche un censimento, sui quali invece si potrebbe fare tanto e si potrebbero sviluppare anche coltivazioni florovivaistiche. Mi dispiace che sia stato dichiarato improcedibile, ma ritengo che sia stato fatto

dove poter impiantare coltivazioni, anche per coinvolgere i ragazzi o i soggetti fragili che vengono avviati a percorsi di recupero e di riabilitazione. Sarebbe stata una bella misura, alla quale mi auguro che comunque, nello sviluppo dei decreti di attuazione, si possa ripensare, trovando il modo per farvi entrare anche questi enti del terzo settore.

previsti nelle deleghe sono anche condivisibili: non vi è dubbio, ad esempio, che sia necessario un piano nazionale del settore florovivaistico come strumento programmatico e strategico.

insufficienti. Noi nutriamo dei dubbi e per questa ragione ci asteniamo su questa proposta. Come dicevo, mentre noi facciamo questa discussione,

manca all'appello, ad esempio, una legge sul blocco del consumo di suolo, laddove ogni giorno migliaia e migliaia di metri quadri vengono cementificati.

il disegno di legge al nostro esame reca una delega che il Governo chiede per poter intervenire su un settore che necessita di essere implementato. Il florovivaismo ha ancora numeri importanti, sia in termini di valore della produzione (3,2 miliardi) sia di numero di imprese (17.000), con 45.000 ettari coltivati e la metà della produzione destinata all'*export.*

che hanno visto un incremento a due cifre rispetto all'anno precedente. Dobbiamo quindi riuscire a cogliere questo momento importante, questo slancio, e a sostenerlo. Serve però una regolamentazione per dare questo ulteriore impulso al settore e per disciplinare più compiutamente l'articolazione delle filiere. Si punta alla riconversione del patrimonio nazionale delle serre in siti agroenergetici attraverso un apposito piano. Le finalità sono quelle di rinnovare le strutture degli impianti esistenti, rendendoli più moderni e più sostenibili dal punto di vista energetico e dell'utilizzo del riscaldamento del riscaldamento e dell'acqua. Ci saranno quindi agevolazioni agli investimenti, per rendere le aziende florovivaistiche italiane più moderne e più in grado di affrontare la concorrenza di un mercato estero che si fa sempre più competitivo. Verranno meglio definite le figure che operano nelle aziende florovivaistiche e attivati percorsi formativi per preparare i lavoratori che faranno crescere le aziende del comparto florovivaistico, a partire dal livello di studio degli si procederà alla ricognizione dei marchi nazionali esistenti, per certificare la qualità del processo produttivo e del prodotto. L'idea è quella di promuovere un marchio unico distintivo del prodotto florovivaistico, riconoscibile nel mondo, che ne certifichi la qualità superiore, in onore di una tradizione e di un'attenzione che abbiamo nel nostro Paese. Peraltro, la definizione del *made in Italy* ha sempre dato questo slancio ulteriore, che dobbiamo consegnare anche a settori diversi da quelli tradizionali. Insomma, si tratta di una serie di deleghe che verranno adottate con l'accordo degli operatori del settore, nei tempi necessari ad approfondire tutte le tematiche e a puntualizzare le forme e i modi degli incentivi. Pertanto, nell'esercizio di queste deleghe ci sarà un coinvolgimento importante degli addetti ai lavori.

I senatori di Forza Italia guardano quindi con grande favore alle norme del presente disegno di legge. Siamo sicuri che alle buone intenzioni seguiranno

Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il florovivaismo ha sempre avuto un ruolo centrale nell'economia agricola nazionale. L'Italia è, nell'Unione europea, uno tra i principali produttori di piante e fiori, vantando una grandissima varietà grazie alle sue diverse caratteristiche territoriali. È necessario ricordare quanto le imprese del florovivaismo siano state messe a dura prova dalle gravi criticità che abbiamo attraversato: prima il difficile periodo della pandemia e poi gli effetti del rincaro dei costi di produzione per i tanti motivi che ormai conosciamo bene, derivanti dalla guerra russo-ucraina. È altrettanto importante ricordare il merito del settore florovivaistico nel contribuire ad attenuare le problematiche climatiche grazie alla forestazione urbana e ai benefici economici e salutistici che ne derivano. Dunque, non ci sono dubbi sul fatto che sia un settore che merita sostegno e attenzione costante. Il Governo, come abbiamo sentito dall'intervento del senatore Patuanelli, nella passata legislatura si è attivato concretamente per il settore, stanziando importanti risorse, poi c'è il *bonus* verde, che continua ad agevolare i cittadini desiderosi di creare spazi verdi. Per un vero aiuto al settore, non si può di nuovo non ricorrere ai fondi del PNRR, che rappresenta, contro ogni smentita, un'opportunità anche per questo settore, attraverso l'investimento per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, con una dotazione complessiva di 330 milioni di euro finalizzati a proteggere le aree verdi e ad aumentarne il numero nelle città metropolitane, sempre più esposte a problemi ambientali come l'inquinamento, la perdita di biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici. Un sostegno mirato alle imprese deriva sempre dai fondi del PNRR, con la dotazione di 500 milioni di euro per lo sviluppo della logistica per gli svariati settori dell'agroalimentare e anche per la floricoltura e il vivaismo, un'opportunità data alla filiera per potenziare i sistemi di stoccaggio, importantissimi al fine di ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi.

un Presidente lontano dai giochi di potere, dalle machiavelliche riforme costituzionali che purtroppo stanno caratterizzando questo Governo e questa maggioranza; un *Premier* che aveva nella mente e nel cuore solo il benessere del popolo italiano e la ripresa veloce dell'Italia; un *Premier* che non si è mai nascosto dietro false candidature per qualche illusorio consenso in più, ma che è andato in Europa solo a fare il suo ruolo. È proprio questo che mi fa riflettere: ciascuno di noi ha un ruolo ed è questa consapevolezza che deve guidarci nel nostro lavoro quotidiano. Siamo parlamentari e abbiamo il ruolo di legislatori: il nostro ruolo, invece, si sta trasformando in quello di ratificatori di decreti, cioè il potere legislativo sta passando costantemente nelle mani di quello esecutivo, del Governo dunque, che emana i decreti-legge. decreti-legge. Questo disegno di legge è una delega quadro: approvato in Consiglio dei ministri a giugno dell'anno scorso, è quindi un decreto già ratificato alla Camera a febbraio e che ora sta per essere approvato approvato qui in Senato, forte dei voti della maggioranza parlamentare, che vedo e sento, ma sembra non rendersi conto di essere stata ridotta a mera passacarte. Un lungo lavoro è stato condotto nella passata legislatura dal Parlamento, quindi da me e dai colleghi di Commissione, così come dev'essere, essendo consapevoli di quanto fosse necessario disciplinare questo settore in continua espansione.

Con questa legislatura e con questa maggioranza il provvedimento però diventa governativo, con il *placet* del Parlamento, che abbiamo visto già dato parere favorevole alla Camera. Dunque il Parlamento concede una delega in bianco, com'è scritto a chiare lettere nell'*incipit* del disegno di legge. All'articolo 1, infatti, è scritto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi - quindi non si sa nemmeno quanti saranno - «per costituire un quadro normativo organico» - si spera - «in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica». Si tratta di una delega a tutti gli effetti,

l'unico stanziamento è quello definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo di livello dirigenziale. Questa è una costante dei vari provvedimenti del Governo: un voler sempre inserire qualche figura dirigenziale, che serva o meno, a dispetto del grande lavoro che viene richiesto agli esperti del tavolo tecnico, che invece sono sempre a titolo gratuito, per un settore che non cerca queste figure da allocare all'ultimo momento. Soprattutto è necessario che ci siano termini più brevi per questo lavoro.

allibisce sempre - l'abbiamo visto anche con il disegno di legge sull'autonomia differenziata - è che poi al Parlamento su questi decreti è dato solo il potere di fare osservazioni, per niente vincolanti,

osservazioni per nulla vincolanti, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti è scritto che il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, quindi anche i futuri correttivi sono lasciati totalmente in mano al Governo. concordi su questo esautorare il potere del Parlamento. Questo è un ennesimo schiaffo che riceviamo noi parlamentari, assolutamente inaccettabile. Di conseguenza,

questo sentirsi inascoltati e non avere forza rispetto a chi ci ha votati, rispetto a chi dal territorio vuole da noi delle risposte.

però il nostro voto non può essere che di astensione. Il MoVimento 5 Stelle si asterrà quindi su questo provvedimento, nel rispetto di una filiera che necessita di una normativa congrua e utile al futuro del settore, affinché questo possa essere ancora un fiore all'occhiello per la nostra Italia.

Come sappiamo bene e come hanno detto anche i colleghi in precedenza, il nostro Paese è in costante crescita in questo settore: nel 2022 erano stati realizzati 3,2 miliardi; poi 3,1 miliardi nel 2023, perché c'è stato un piccolo calo, però la tendenza dei primi mesi di quest'anno è già molto in crescita.

In Europa, l'Italia è seconda solo ai Paesi Bassi per esportazione di piante e fiori, con oltre 1,2 miliardi di vendite nel 2023, mentre nei primi quattro mesi del 2024 c'è già un 4,5 per più. Siamo il terzo esportatore mondiale nel settore, addirittura al primo posto in alcuni segmenti del florovivaismo. Rappresentiamo quindi una vera e propria eccellenza, ma anche un pilastro per la rigenerazione urbana e il paesaggio, la cultura del bello e del fare, attraverso coloro che producono nel nostro Paese. È un settore straordinario e importante. I risultati raggiunti ci spingono a rafforzare l'impegno delle istituzioni nei confronti di questa filiera. Con il disegno di legge in materia di florovivaismo il Governo si è dato l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo, puntando in particolare su ricerca e innovazione tecnologica, coniugando il tema della il tema della produzione e del rispetto dell'ambiente. Ricordo però che la proposta di legge abbinata al provvedimento che oggi esaminiamo in Aula è originariamente a firma a firma del Gruppo Lega - lo sa bene anche il Sottosegretario, che ringrazio per il suo impegno - e scaturisce da un importante lavoro svolto, sempre nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati su questo tema. tema. Ci sono voluti alcuni anni, ma siamo arrivati alla fine. Si tratta di un provvedimento necessario, perché va a normare un settore che chiede di essere ascoltato e sostenuto in modo cogente perché strategico, come abbiamo detto, per il *made in Italy* e per l'agricoltura italiana. recepisce le esigenze della categoria, consente di avviare una ricognizione approfondita del comparto, che fino ad oggi non era regolamentato in modo adeguato e che ha necessità di una legge che possa favorire lo sviluppo e difenderlo soprattutto dalla concorrenza straniera, qualificare gli operatori che hanno continuato ad operare nonostante le grandissime difficoltà. Il florovivaismo è un'attività complessa e un settore caratterizzato da un'elevatissima competitività e specializzazione. Non mancano le problematiche, a cominciare da quello che è stato il post-pandemia, che hanno colpito con forza il florovivaismo. Ci sono piccole aziende che hanno subito l'azzeramento totale del fatturato, problema è stato scongiurato grazie ad alcune misure che ricordava prima anche il già ministro Patuanelli, nonché grazie soprattutto alla determinazione degli imprenditori. Infatti, da sempre è segno distintivo dell'imprenditoria italiana il rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Grazie a queste aziende dobbiamo dire che molti territori, anche marginali, continuano a sopravvivere e ad avere occupazione: se non ci fossero queste imprese, mancherebbero l'occupazione in quelle aree e soprattutto il presidio del territorio. Le aziende italiane devono poi fronteggiare la concorrenza sleale dall'estero. Noi siamo le vittime mondiali dell'*italian sounding*, legato al prezzo e non basato sulla qualità.

e con regolamenti e leggi in materia completamente diversi. Occorre quindi intervenire per dare al settore, come abbiamo detto, la capacità di riprendersi con la continua evoluzione (ci sono le cultivar), l'adeguamento tecnologico, con l'innovazione e una particolare attenzione alle imprese e agli investimenti. Tra i punti su cui è fondamentale focalizzarsi c'è il sostegno agli eventi fieristici legati al florovivaismo, allo scopo di favorire sempre più l'incontro tra domanda e offerta del nostro straordinario prodotto. Questo va nell'ottica di sviluppare sempre di più un *export* forte, nonché la necessità di perseguire nuove politiche di tutela del marchio italiano, la cui unicità risiede nelle peculiarità dei singoli territori e nelle modalità tradizionali di lavorazione, perché ciò è fondamentale. Ricordo a tutti che l'Italia è sede delle due più importanti manifestazioni florovivaistiche internazionali. Abbiamo Euroflora, che si svolge a Genova ed è biennale - sarà

La legge sul *made in Italy*, infatti, per agganciarci a questo tema, prevede uno stanziamento per lo sviluppo del settore fieristico e un fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per il 2023 di 300 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzati al sostegno, alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali. Qui entriamo in gioco anche col florovivaismo. Il testo in esame si inserisce in questo contesto come elemento principale nella stesura di un piano nazionale, concertato con gli operatori, con le organizzazioni del settore, ma soprattutto con le Regioni; la ricognizione dei marchi nazionali e la promozione di un unico marchio distintivo, che ci renda riconoscibili non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Noi abbiamo di fronte una sfida importante che dobbiamo affrontare se davvero intendiamo valorizzare questo settore per riuscire a riqualificarlo. Con i decreti legislativi si riuscirà a regolamentare un settore difficile che richiede regole certe; si dovranno disciplinare i centri di giardinaggio all'interno della filiera agricola e la formazione professionale, per qualificare e migliorare le produzioni estese. Ci sarà la possibilità di avvalersi di investimenti in innovazione, che permetteranno al settore di progredire e di essere sempre più competitivo. Vi è poi il posizionamento della logistica nazionale, che diventerà strategico per il futuro del nostro Paese. Tra le misure previste c'è anche la promozione di coltivazioni a bassissimo impatto ambientale e si andrà nella direzione della *green economy*, ma non quella integralista e inconsistente che chiede l'Europa, ma quella che ci permette di produrre e di essere comunque competitivi dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Noi, come Lega, chiederemo sempre risposte concrete, le stesse che sta dando il Governo in questo periodo,

per valorizzare sempre di più il settore. Sono previsti anche un piano programmatico del settore di durata quinquennale, la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati e la creazione

perché diventa importante anche il tema delle pratiche sleali, soprattutto nella vendita e nella competitività di questi prodotti. Alla luce di tutto questo, esprimiamo con convinzione il voto favorevole al provvedimento abbiamo detto - per la coltivazione, la promozione, la commercializzazione, la valorizzazione e l'incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti. Noi compiamo un atto di fede verso il Governo, qui rappresentato dal sempre disponibile e competente sottosegretario La Pietra, per una immediata emanazione - e lui lo sa bene - dei decreti, che sono indispensabili per far sì che questo provvedimento entri in vigore e aiuti realmente e concretamente la filiera, com'è

detto anche i miei colleghi precedentemente - per cui noi la leggiamo, anche alla luce delle parole del Sottosegretario, non come un atto di intento, ma come un atto reale. La sfida vera saranno i decreti, le norme attuative, i decreti legislativi e quant'altro, che dovranno dare risposte a un settore che da molti anni le imprese rivendicano come centrale e che è centrale per il nostro Paese, è centrale per le nostre pubbliche amministrazioni, è centrale per i nostri cittadini. Stiamo comunque parlando del settore florovivaistico, che rappresenta un elemento identitario per il nostro Paese e per alcune Regioni, come la mia (la Toscana) e tante altre, da salvaguardare. È chiaro che non entro nei numeri, perché sono stati ampiamente ribaditi anche per la loro importanza.

Il Governo si è insediato da due anni e oggi noi ci troviamo a dare una prima risposta, ma gli imprenditori non hanno tutto questo tempo a disposizione prima di vedere risultati o le loro istanze tradotte in norme applicative. Per quanto riguarda i decreti legislativi, la prendiamo in parola, Sottosegretario, sul fatto che lei si è impegnato ad attivare i tavoli tecnici con rapidità per dare delle prime risposte. un percorso per arrivare a una definizione strutturale del settore del florovivaismo, che dovrebbe riguardare però tutto il tema dell'agricoltura. Se in agricoltura noi seguiamo le emergenze, non ce la faremo mai a raggiungere quei livelli necessari al sistema produttivo e alla strategicità dello stesso. pratica, i nostri atti troppo spesso parlano di ristori - ristoro alle pere, ai kiwi, per il problema del granchio blu o della xylella e quant'altro

il danno su vasta scala derivi da una carenza di monitoraggio e di contenimento nella fase iniziale, per cui è necessario che siano investite risorse ministeriali e che siano proceduralizzate alcune forme di monitoraggio.

Accanto al monitoraggio è chiaro che ci vogliono ristori quando questo avviene. Ma ci vuole anche una politica di lungo periodo, perché in agricoltura - come spesso diciamo - tra quando si pianta un insieme a quando l'albero diventa adulto e può essere venduto dal vivaista, non passano mesi non passano mesi o semestri, passano anni, per cui ci vuole una programmazione strutturale. Credo anche che sia arrivato il tempo per mettere le radici a un testo unico sull'agricoltura, che abbia una visione di lunghissimo periodo. Capisco che queste sono quelle cose che non si riesce a portare a termine in una legislatura,

norme, attuazioni e risoluzioni dei problemi, consegna al Paese una strategia per il futuro, una pietra su cui mettere altre pietre per poi costruire una casa per un settore come quello agricolo che una fondamentale esigenza. Tutti noi abbiamo fatto campagna elettorale in questo periodo e tutti noi abbiamo fatto gli incontri con le categorie. Il grido d'allarme più forte che emerge

In tutti i provvedimenti - e lo sto dicendo dal primo giorno - non vediamo una norma sull'infrastrutturazione digitale delle aree interne, che sono di per sé svantaggiate e presentano problematiche significative in termini di logistica, di trasporti, di accesso ai servizi e quanto altro. Dobbiamo dare a quelle aree, quantomeno, la possibilità di portare le piccole produzioni, le produzioni di nicchia, a competere sul mercato; bisogna dare la possibilità di accedere alla pubblica amministrazione in forma digitale. forma digitale. Anche nel decreto agricoltura che stiamo esaminando in questi giorni non c'è una norma sull'infrastrutturazione digitale delle aree interne. Questo è necessario, perché ormai le aziende hanno bisogno di essere al passo con i tempi e la digitalizzazione, anche per l'accesso alle pratiche, è essenziale. Nonostante tutte le problematiche che abbiamo rilevato, riteniamo di dover esprimere un voto favorevole, pensando alle imprese che da troppo tempo stanno aspettando questa normativa. Ma lo facciamo - così come detto dai miei colleghi della Camera

non sarà questa norma a dare una soluzione al tema del florovivaismo, ma saranno i decreti legislativi e le norme attuative che dovranno essere emanate. Diversamente rischia di essere l'ennesima l'ennesima norma-scatola che non avrà contenuti. Il Paese e gli agricoltori non se lo possono permettere e hanno bisogno di risposte, in un momento estremamente difficile e delicato come quello attuale, in cui devono fare i conti con il mercato, con le crisi internazionali, ma soprattutto con i cambiamenti climatici, che non sono più un episodio o un fatto sporadico. Non passa settimana, non passa giorno senza che in una parte di questo Paese avvenga un fatto straordinario e imprevisto. Questo ci deve portare a riflettere sul fatto

creato aspettative per una sfida, affinché un settore così importante per il PIL italiano e per l'agricoltura italiana abbia,

vedere il settore florovivaistico come uno di massima importanza, con regole certe, considerandolo come un insieme nazionale e non solo zonale, ossia di varie zone dell'Italia interessate in modo specifico al florovivaismo, e uno su cui l'agricoltura italiana e il Governo intendono puntare. Faccio l'esempio della mia Regione, la Liguria, dove il florovivaismo vale quasi mezzo miliardo di PIL prodotto e dove ha un impegno di manodopera importantissima, anche se impiegata in piccolissime aziende. Proprio da questo nasce l'interesse nazionale ad avere una legislatura *ad hoc,* dedicata, che possa far sì che il nostro insieme delle aziende florovivaistiche possa dare il meglio e massimizzare l'impegno a sostegno della filiera e dell'economia nazionale.

del Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico. Molte volte abbiamo visto come la mancanza di strategicità del settore e di un indirizzo pluriennale, in questo caso quinquennale, abbia sfavorito le nostre aziende, lasciando magari ai singoli imprenditori scelte fatte da sé, senza avere un quadro nazionale in cui scegliere e senza essere consigliati e supportati nel migliore dei modi nella direzione da intraprendere per raggiungere l'obiettivo. La lettera *f)* prevede che il citato piano individui azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione tecnologica e alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale. ci sono molte cose, a cominciare dalla formazione professionale in un campo dove non sempre essa è presente o dove non sempre ad essa viene data la giusta importanza. Penso che nei decreti legislativi tornare sulla formazione professionale, indicando le qualifiche che è meglio formare affinché il settore progredisca, sia molto importante.

che daranno la certezza di come, di cinque anni in cinque anni, questo settore importantissimo a livello regionale e nazionale potrà progredire. La lettera *g)* prevede che il piano individui azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti. Spessissimo - e rifaccio l'esempio della mia Regione - abbiamo prodotti di grande eccellenza che negli anni non siamo riusciti a promuovere davanti a un mercato mondiale molto aggressivo. che accentrare a livello nazionale l'aiuto alla promozione, dando consigli, linee di indirizzo e aiuti a promuovere il prodotto locale che diventa eccellenza nazionale sia importantissimo, soprattutto in un settore che molto spesso è fatto di piccole e piccolissime aziende. Ci sono le grandi e le grandissime aziende, ma ci sono anche piccole e piccolissime aziende che hanno necessità di essere supportate anche nella promozione del loro prodotto. Immagino che promozionare un prodotto a livello nazionale sia molto più incisivo in un mercato globale come questo, rispetto a quello che può fare una piccola azienda, oppure aziende di piccole zone rispetto al panorama nazionale di produzione.

competere sul mercato nazionale e internazionale per mancanza di logistica comune. È complicato spedire all'estero i fiori e le piante in vaso: è complicato se non si ha un sistema coordinato

dove il prodotto viene commercializzato crescano e si ammodernizzino in termini di logistica. Questo, insieme a quegli interventi, sarà di grande aiuto alle nostre aziende, soprattutto in prospettiva. Il punto *l),* dal punto di vista dell'ambiente importantissimo, reca la misura per la riconversione degli impianti serricoli destinati al florovivaismo in siti agroenergetici. Nella mia Regione, come in altre, ci sono ettari di serre non più utilizzati, che non si sa come utilizzare perché costa lo smontaggio e costa la riconversione. Questo punto, una volta trasformato in un decreto legislativo, potrà aiutare molto a utilizzare quelle serre senza doverle smantellare o a trasformarle in siti

Molte volte nelle nostre aziende mancano le figure professionali, ma manca anche la figura professionale giuridicamente individuata per far sì che la persona venga assunta per fare quel lavoro e con la qualificazione corretta per svolgere il lavoro. Penso che, in questo caso, l'impegno del Governo sarà notevole e produrrà risultati che permetteranno agli imprenditori, da una parte, e ai lavoratori, dall'altra, di avere la giusta qualificazione al momento dell'assunzione e a far sì che le competenze all'interno delle aziende siano rispettate, ma da subito e in maniera corretta. prevede la promozione e l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy. Ciò servirà a creare persone formate sì, ma servirà anche a promuovere la professione del florovivaista, declinata in tutte le qualifiche che servono all'intorno di un vivaio e di una coltivazione. Promuoverà presso i giovani l'amore per un lavoro che è servito a far sì che l'Italia progredisse, che nei secoli ha cambiato molte volte in meglio la morfologia del nostro territorio, facendo sì che fosse adeguato alle piantagioni, in questo caso floricole o florovivaistiche, che in quella realtà erano migliori, come è successo nella mia Regione. Penso, pertanto, che vi siano elementi sufficienti per dire un sì convinto a nome del Gruppo Fratelli d'Italia a questo disegno di legge.

Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza. Intendo esprimere sincere parole di solidarietà alla collega senatrice Ester Mieli, perché l'intero Paese è sconvolto da quanto emerso dall'inchiesta giornalistica condotta da «Fanpage»a proposito di

alla visione di tutti sono inoppugnabili. Mi sento quindi di suggerire, davvero sinceramente, agli esponenti di quel partito di prendere nettamente le distanze da quegli atteggiamenti, da quei comportamenti, da quei saluti fascisti, da quelle parole che abbiamo visto tutti scritte nelle *chat* e che sono irripetibili,

Prendete le distanze non da «Fanpage», bensì da quei circoli e da quelle persone che esprimono comportamenti incostituzionali, in violazione di di tutti i diritti umani, e che inneggiano a periodi della nostra storia che devono essere lasciati nel buio a cui appartengono.

massima e totale del Gruppo Partito Democratico e dell'intero Partito Democratico alla senatrice Mieli. Vorrei però approfittare di questo intervento per chiedere davvero al presidente Malan e al Gruppo che rappresenta di utilizzare il tempo che abbiamo davanti,

da persone che rappresentano il popolo italiano e difendono l'istituzione che serviamo, una Repubblica profondamente antifascista, il dovere che abbiamo - senatore Malan - è allontanare tutti coloro che fanno regredire culturalmente il nostro Paese e alimentano un conflitto di cui non c'è bisogno. Le garantiamo il Partito Democratico sarà sempre dalla parte della coesione nazionale, ma la coesione nazionale e l'unità nazionale non le si coltivano se non allontaniamo persone che alimentano lo scontro politico, alimentando la cultura fascista. Prendete le distanze, per favore, perché la cultura fascista è ancora presente dentro alcune forze politiche. Noi pensavamo di dover combattere Forza Nuova e CasaPound, non Gioventù Nazionale. Siccome è parte integrante della vostra forza politica, non dobbiamo dirvi noi cosa dovete fare: avete l'obbligo morale di prendere delle decisioni. dell'onorevole Donzelli: non ci bastano, e non solo perché offendono la nostra collega, ma anche perché non possono essere le parole di chi guida o coordina un partito che ha la responsabilità di Governo. Questo è un Paese profondamente antifascista e ai giovani di oggi dobbiamo dire che quella roba lì non appartiene alle istituzioni della Repubblica, la combattiamo ed è distante anni luce dalle modalità con le quali vogliamo costruire il futuro del nostro Paese.

una cultura che si alimenta anche di molti silenzi e noi non vogliamo più restare in silenzio. Vi chiediamo quindi di non restare in silenzio, di essere conseguenti e di prendere le distanze. Sappiamo che potete farlo. Purtroppo Purtroppo non lo avete ancora fatto e siete alla guida del Paese da venti mesi. Ed è questo il motivo che ci porta a essere emarginati anche in Europa. *(Applausi)*. rigorosamente sull'ordine dei lavori, intanto per un'annotazione personale: faccio parte della Commissione antidiscriminazioni, della quale la senatrice Mieli è Vice Presidente, e ho apprezzato, nel corso dei lavori di questa Commissione, che ha ovviamente il Presidente più illustre di quest'Aula, Liliana Segre, l'equilibrio, le capacità anche - direi - l'assoluta visione d'insieme che la senatrice Mieli ha sempre dimostrato. Questa mattina, a nome del Gruppo Italia Viva, ho pubblicato un *tweet* proprio per dimostrare la nostra solidarietà nei confronti della senatrice e ricordare il lavoro prezioso che lei ha fatto per tutti noi. Credo che sia questo, prima di tutto, l'oggetto della richiesta di intervento sull'ordine dei lavori, cioè dire a tutti che la senatrice Mieli è stata preziosissima in una battaglia contro le discriminazioni e in una battaglia contro l'antisemitismo che questa Assemblea rivendica a pieno titolo e lo deve fare in ogni direzione e in ogni parte politica. Certo, senatrice, è del tutto evidente che, nel cogliere questa occasione, chiediamo anche che questa battaglia, questa puntualizzazione venga fatta anche dalla sua parte politica, non tanto perché in questo momento sia importante sbattere in faccia al vostro partito politico una qualche recriminazione rispetto a logiche che penso vi siano distanti, ma perché la consapevolezza e la presa di posizione collettiva in questo momento è solo l'aiuto migliore a ogni rigurgito antisemita che c'è in Europa e anche in questo Paese. Quello che vi chiediamo è di alzare la voce, perché questa voce è importante per la nostra democrazia ed è importante per l'autorevolezza di queste istituzioni. La ringrazio per quello che ha fatto. Le porgiamo davvero la nostra vicinanza e le chiediamo di continuare a svolgere con lo stesso coraggio e con la stessa determinazione una battaglia che noi condividiamo con lei e che penso che tutta l'Aula debba condividere in nome della democrazia e di una logica di civiltà reciproca.

esprimendo ovviamente la nostra solidarietà come Gruppo alla collega, ma allo stesso tempo vorrei sottolineare quanto detto pocanzi dalla senatrice Paita. In sostanza, nel nostro Paese c'è un rigurgito antisemita e nello stesso tempo di

La democrazia la si difende sostanzialmente con i valori democratici e, quindi, bisogna condannare incondizionatamente tutte le organizzazioni neonaziste e neofasciste e, nello stesso tempo, sarebbe necessario procedere anche allo scioglimento di alcuni raggruppamenti.

particolarmente orgoglioso, anzi tutti noi senatori di Fratelli d'Italia siamo orgogliosi di avere Ester Mieli come nostra autorevole collega e di aver indicato il suo nome e averla votata insieme alla maggioranza per il posto di Vice Presidente della Commissione antidiscriminazioni. Direi che oggi, alla luce di quanto è emerso, questa scelta è particolarmente felice. Noi non ci riconosciamo nelle espressioni e nei gesti inaccettabili che sono emersi in quei video, peraltro carpiti in modi come minimo ampiamente discutibili, ma non è questo ora il punto. Non ci riconosciamo in quegli atti e in quei gesti perché i nostri principi sono nella libertà, nella democrazia, nella condanna di ogni totalitarismo, totale condanna di ogni forma di razzismo e di antisemitismo.

la colpisce personalmente. Auspico che un atteggiamento simile sia tenuto sempre da tutti, perché già due anni fa, quando si stavano presentando le candidature, emersero delle dichiarazioni estremamente imbarazzanti di candidati o di candidabili di altri partiti. Qualcuno è stato ritirato, qualche altro è rimasto. Non è questo l'argomento di oggi, ma lo ricordo. Ricordo che ci sono alcuni che sono stati tolti dalle liste e altri che sono rimasti nelle liste e sono stati pure eletti in Parlamento. Questo non cambia, perché noi dobbiamo pensare a quello che succede nell'ambito del nostro partito, senza dubbio; ma a livello generale, visto che qui parliamo ovviamente a livello generale, ci tengo

Al di là delle motivazioni, che rientrano anche in un ambito di contrasto politico, ma tale solidarietà noi apprezziamo profondamente e riteniamo che ogni provvedimento, ogni seguito debba essere all'altezza del nostro del nostro atteggiamento personale, politico, valoriale e di principi che abbiamo nei confronti di Ester Mieli. Confesso - non me ne voglia Ester - di essere sempre stato un po' innamorato di lei, sicuramente perché è bella e soprattutto perché esprime sogni, speranze, se vogliamo rabbia, con enorme garbo, sempre

quello che conta veramente: le pari opportunità, le pari dignità. Quindi mi associo,

apprezzando totalmente l'intervento del presidente Malan, il discorso della cultura fascista. Non ci sto, Non ci sto, anche perché mi sento toccato profondamente da quello che è stato detto contro le persone con sindrome di Down. Non esiste una cultura fascista: esiste una malattia mentale fascista, che va curata, perseguita e contrastata con ogni mezzo democratico. Io non mi sento offeso perché sono stati colpiti i valori della disabilità. Parlo di valori, sì, perché sento di rappresentare un mondo di grande voglia di vivere, di superare le difficoltà, di essere contro le discriminazioni legate alle diversità. Sono orgoglioso di essere disabile, anche se qualche volta mi dico che vorrei tornare a correre, a giocare a padel, ad esprimermi anche con il corpo in maniera diversa, ma sono felicissimo di stare qui e di rappresentare questo mondo, magari in maniera limitata, al Senato, nella Camera alta. Credo quindi che non dobbiamo usare contro qualcuno cose che non esistono: non c'è una cultura fascista, ma c'è una malattia mentale che va curata, che va perseguita, che va giudicata male, ma non va usata contro chi, se permettete, fa il proprio lavoro anche e soprattutto nel centrodestra, anche e soprattutto in Fratelli d'Italia. Non mi sento in colpa per essere nel partito di Giorgia Meloni, anzi sono orgoglioso della dignità che porta nel far politica. Una considerazione e mi taccio. Ma guarda un po', proprio oggi che il Presidente del Consiglio, non solo il capo di Fratelli d'Italia, in Europa a rappresentare tutti, esce qualcosa a tempo. Questo mi ricorda, pur essendo totalmente d'accordo sulla libertà di stampa, certi giudizi a tempo in campagna elettorale quando succede qualcosa di critico. Credo quindi che prima di tutto, deprecando la malattia mentale fascista che qualche sciocco o sciocca anche in maniera rozza esprimono, come deprechiamo la malattia mentale del fascismo o peggio del nazismo con le sue leggi razziali che sicuramente sono il lato più oscuro del secolo breve, del successivo e di quello che potrà dobbiamo esprimere totalmente il sostegno al Presidente del Consiglio che, con tanta dignità, intelligenza e, se vogliamo, generosità, si esprime per tutti noi. Grazie a voi tutti, grazie a Ester, grazie a Giorgia e, se volete, grazie a Catia,

femminilità. Quando la mattina chiama, si ricorda di dire prima di tutto «come state» e poi si lamenterà qualche volta per dire «come sto». Ecco come sono le persone con la sindrome di quelle che amano in modo infinito; forse sarà una fregatura, ma soprattutto ci danno un esempio di come bisogna, con lentezza, gustarsi la vita e accettare gli altri. È un esempio su cui forse dovremmo

brevemente per unirmi alle parole espresse da tutti i colleghi, Grazie a tutto Basta guardarla in viso, basta guardare il suo volto per capire la sofferenza che sta provando. Credo che oggi sia una giornata importante perché abbiamo dimostrato ancora una volta la vicinanza: siamo con lei. Non è la prima volta che viene attaccata attaccata e che finisce sotto i riflettori. Quindi forza Ester, siamo con te, un forte abbraccio. a nome della Presidenza per il lavoro e la lotta continua che fa contro l'antisemitismo, che è la lotta di tutti noi, così come di tutti noi è l'impegno a difendere i valori democratici della nostra Costituzione, che è una Costituzione antifascista che combatte qualsiasi forma di nostalgia o apologia del fascismo e di ogni altro autoritarismo. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*. *(La seduta, sospesa

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'università e della ricerca.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro, in questi giorni da circa una settimana tutta l'Italia è coinvolta per la vicenda, del lavoratore Satnam Singh, un lavoratore che è andato incontro a una morte tragica, brutale, una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica perché questo lavoratore era un cosiddetto invisibile, un lavoratore che lavorava per circa 3 euro di paga l'ora per oltre dieci ore di lavoro in un'azienda dell'Agro Pontino,

non ci sia offesa in queste parole, ma è proprio la descrizione di ciò che è avvenuto - davanti alla sua abitazione, abbandonandolo lì. Il lavoratore poi è morto. Satnam Singh è morto, e la cosa ancora più aberrante e che se fosse stato soccorso tempestivamente da personale medico, si sarebbe salvato. Quindi questo è lo scenario davanti al quale ci siamo trovati in quest'ultima settimana che ci ha lasciato tutti inorriditi. Però non possiamo dire che ci abbia lasciato sorpresi. Non possiamo dire sorpresi, signor Ministro, perché purtroppo questo è un fenomeno noto, è un fenomeno conosciuto, è un fenomeno contro il quale già ci sono degli strumenti di intervento. Ci sono delle normative specifiche, ci sono delle somme che sono state stanziate, ma evidentemente è un fenomeno che si lascia nel sommerso, che non si vuole affrontare. Dico questo perché già la legge di contrasto al caporalato prevede

al fondo e al progetto; trascorsi i sessanta giorni, non soltanto la nomina del commissario è stata fatta tardivamente, ma è stata fatta da parte del Ministro dell'interno, invece che del Ministro competente, ed è stato nominato il prefetto di Latina, che ovviamente è persona rispettabilissima e onorabilissima, ma è un prefetto, cioè all'interno della Prefettura

con misure per eseguire effettivamente i controlli e dare attuazione alle leggi e applicare anche le sanzioni, o vogliamo continuare a stare dietro a una retorica che non soddisfa nessuno e soprattutto non tutela questi lavoratori?

la collega per aver posto questo quesito insieme ad altri che ne seguiranno di tono simile, ai quali proveremo a rispondere in modo coordinato. Quella del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in particolare in agricoltura sono questioni a cui teniamo molto e che, come è stato ricordato, emergono non da oggi, ma da qualche decennio. Il tragico evento occorso in Provincia di Latina, in cui ha perso la vita il trentunenne Satnam Singh - esprimo ancora una volta a nome del Governo il cordoglio, alla sua comunità e alla sua famiglia ed in particolare alla moglie - richiama però oggi l'urgenza del pieno rispetto delle regole e della stringente tutela dei diritti, continuando a intervenire affinché questi episodi criminali non trovino più spazio nel nostro sistema agricolo, costituito da una generalità di imprese serie, che agiscono nel rispetto della legge. Sin dal suo insediamento, il Governo Meloni ha operato in questa direzione, mettendo in campo una pluralità di azioni nei diversi ambiti lavorativi e su tutto il territorio nazionale, sulla base degli specifici contesti territoriali. Siamo intervenuti con il massimo impegno, in stretta collaborazione con gli altri Ministeri competenti, sulle diverse e complesse questioni legate al tema del lavoro agricolo irregolare e contro ogni forma di sfruttamento, nel quadro di una piena attuazione della legge e del piano di contrasto al caporalato, tanto sul fronte della repressione che della prevenzione. Tutti temi che, almeno sul piano dell'efficacia, non trattati adeguatamente dai Governi precedenti. Ricordo infatti la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS nel lontano 2014, sulla quale sono emerse numerose esigenze di riforma: uno strumento che si è dimostrato inefficace, oppure, se vogliamo guardare i numeri, fallimentare, come testimonia la scarsa adesione delle aziende agricole, che è stata costante in tutti i dieci anni di attività dei Governi che ci hanno preceduto. Vorrei inoltre ricordare all'interrogante che proprio il Governo presieduto da Matteo Renzi operò una depenalizzazione, che io considero sciagurata, del reato di somministrazione illecita di manodopera, con decreto legislativo n. 8 del 2016, i cui effetti devastanti hanno portato, solo nei primi due anni, ad un incremento di questo genere di violazione di circa il 39 per cento. È solo grazie al Governo Meloni che il reato di somministrazione illecita è stato finalmente reintrodotto. alimentare e delle foreste, in uno dei miei primi provvedimenti ho dato avvio alla condizionalità sociale, misura che vincola oggi i contributi della politica agricola comune (PAC) alla sicurezza lavorativa e al rispetto delle normative sui contratti di lavoro. L'introduzione di specifiche misure sanzionatorie, con l'innalzamento delle percentuali di riduzione degli aiuti e la previsione del meccanismo di sospensione immediata della PAC in caso di procedimenti penali per il reato di caporalato, oltre all'inasprimento dei provvedimenti in caso di recidiva (decreto legislativo 188 del 2023), sono la dimostrazione concreta della volontà di intervenire in modo mirato per contrastare il fenomeno. Un altro fronte cardine di intervento è quello della gestione legata ai flussi migratori. La programmazione su base triennale dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri - novità introdotta con il decreto Cutro - ha l'obiettivo di rendere la gestione funzionale alle esigenze delle imprese italiane e alla carenza di manodopera stagionale, traducendo il fabbisogno in lavoro qualificato e istanze di lavoro dignitoso, anche attraverso l'azione delle organizzazioni di categoria. Lo scorso giugno, ben prima dell'incidente avvenuto a Cisterna di Latina, abbiamo proposto modifiche ulteriori al decreto flussi per il superamento del *click day* legato alla verifica della congruità numerica, passando ad un aggiornamento procedurale del meccanismo di incontro tra la domanda e l'offerta. Con la nomina del commissario a cui ha fatto riferimento, il commissario prefetto Maurizio Falco, attuata dall'Esecutivo su indicazione del ministro Piantedosi, così come la legge prevede, abbiamo rafforzato l'impegno rivolto al superamento degli insediamenti abusivi, al maggior contrasto delle condizioni di sfruttamento e al controllo delle infiltrazioni della criminalità organizzata. A questo si aggiunge un'azione mirata di intervento avviata anche nel contesto del PNRR. Alla misura relativa agli *standard* abitativi per i lavoratori agricoli e di competenza del Ministero del lavoro si affiancano quelle gestite dal Ministero dell'agricoltura in materia di sicurezza e produttività, con l'intervento sulla meccanizzazione e l'equa distribuzione del valore tra gli operatori tramite i contratti di filiera. Per salvaguardare le produzioni agroalimentari di qualità e rendere sistematica l'azione di vigilanza all'interno della filiera agroalimentare, abbiamo previsto l'istituzione della specifica cabina di regia a cui partecipano l'Ispettorato antifrode del Ministero dell'agricoltura, i Carabinieri del CUFAA, la Guardia di finanza, le Capitanerie di porto, l'AGEA e l'Agenzia delle dogane. L'obiettivo è coordinare i diversi piani di intervento nella direzione di una maggiore efficacia dei controlli, della garanzia del giusto prezzo e del pieno contrasto alla concorrenza sleale in agricoltura, che svilisce la qualità del lavoro e favorisce il caporalato. In questo ambito stiamo provvedendo ad introdurre ulteriori e specifici interventi in sede di conversione del decreto agricoltura, che istituiscono un sistema informativo di condivisione e scambio dati per lo sviluppo di strategie di contrasto al caporalato. Questo complesso di azioni è una testimonianza del costante impegno del Governo in carica da venti mesi - un po' meno di quelli in cui si rappresentano una questione e una criticità legate al lavoro sommerso mantenendo fermi la centralità dell'uomo e il suo rapporto con un lavoro che deve essere sempre dignitoso e garante di condizioni di benessere per il lavoratore e la propria famiglia sul territorio di questa Nazione. Signor Presidente, devo dire che quando mi sono preparata per questo *question time* non avrei mai immaginato di sentire il ministro Lollobrigida venire qui a raccontare una bugia grossa come una casa piuttosto che affermare le responsabilità del Governo e soprattutto dire che cosa vuole fare per cercare di contrastare il caporalato. Ministro, l'unico Governo che ha attuato una vera

ha reso applicabile anche nell'ambito della verifica sul sistema di sfruttamento, quindi oggi non è più necessario dimostrare il tema delle percosse, per esempio, perché basta lo sfruttamento per ricadere in questa fattispecie. Quindi il Governo Renzi ha lavorato sia nell'ambito della prevenzione che nell'ambito dei flussi. Questa bugia che lei ha detto l'aveva già detta la presidente ha trovato scarso accoglimento anche nell'opinione pubblica perché è talmente falsa che ripeterla in questo contesto in occasione della morte di Satnam Singh è veramente deplorevole. Che cosa

per avere gli ispettori e soprattutto indicare una strategia per superare quei ghetti e quelli alloggi che sono indecenti per le persone, che voi non avete fatto. Le dirò di più, caro Ministro: non c'è solo la responsabilità del Governo, ma c'è anche la responsabilità dell'amministrazione comunale della quale voi siete la maggioranza; quindi ci sono due responsabilità enormi su questo punto. Il tema che lei oggi ci pone è è non avere una strategia nell'ambito delle risorse, perché non avete detto - e lei nella risposta non ha indicato - come volete affrontare il tema dei controlli. Con il tema dei controlli si risolve la questione del caporalato: esattamente ciò che la ministra Bellanova, forte anche della sua esperienza personale, aveva scritto su quella legge che è patrimonio di tutti e che purtroppo non può trovare attuazione, se non ci sono le risorse sufficienti. Avrebbe dovuto dare una spiegazione su questo, ma ha provato a buttare la palla in tribuna. Ciò che è grave è che lei prova a buttare la palla in tribuna di fronte a una morte, di fronte a un decesso, di fronte a un dramma sul quale ci vorrebbero un po' più di responsabilità e forse un po' più di misura istituzionale. Ma capisco che chi non ce le ha non se le può dare.

Signora Presidente, colleghi, ringrazio il ministro Lollobrigida per essere qui oggi a rispondere alle nostre interrogazioni. Anch'io seguo la scia della collega nel menzionare l'evento orribile che ha segnato le nostre cronache, nel menzionare il bracciante agricolo Satnam Singh, che da oggi non sarà più invisibile, dopo essere stato considerato tale e soprattutto dopo essere stato trattato malissimo, fino al punto da essere abbandonato senza possibilità di salvezza, senza possibilità di avere di avere un servizio sanitario a disposizione. Qui si parla dei bisogni essenziali dell'uomo e si arriva a toccare il fondo. Sicuramente questo incidente ha portato a galla una situazione terribile, e questa essere l'ultima volta che ne parliamo e anzi sono felice di continuare a parlare di lui, sono felice che si possa adesso accendere un faro che non sia la solita pantomima. Mi auguro che si riesca a capire quali

l'ANCI ha denunciato che verranno persi per una mancata attenzione di questo Governo e dei Comuni con una maggioranza del vostro colore politico. La vostra responsabilità è grande. Auspico che ci sia un intervento immediato che riesca a far rete tra le associazioni di categoria. Tutti devono convergere su questo obiettivo, che è la condizionalità che la PAC ci detta a livello europeo. Noi abbiamo il dovere di rispondere a livello italiano e il dovere di essere uniti. La mia interrogazione vuole proprio andare su quelle che sono le sue competenze. Mi rendo conto che è necessaria una sinergia tra i vari Ministeri,

foreste*. Senatrice Naturale, come ho già detto, oggi abbiamo una serie di *question time* su un argomento importante, che riguarda il caporalato e in particolare la perdita di un lavoratore, che è lavoratore al di là della sua provenienza. Colgo però l'occasione, visto che sono stati chiamati in ballo i sindaci, per dire che non so se il sindaco di Cisterna di Latina abbia delle responsabilità. Vorrei correggere però la collega Paita, perché l'amministrazione di Cisterna di Latina è governata dal centrosinistra e, quindi, la responsabilità da imputare al centrodestra rispetto a questo è un po' complessa. Le farà piacere sapere, senatrice Naturale, che anche il vostro partito fa parte di questa amministrazione. Ho tenuto a precisarlo, perché è utile. Sin dall'insediamento di questo Governo, il Ministero che ho la responsabilità di guidare si sta impegnando per sviluppare il settore agricolo. La crescita del comparto non può prescindere da un miglioramento generale delle condizioni di lavoro, sia dei titolari di aziende agricole che dei dipendenti, ivi compresi quelli stagionali. Credo infatti che l'equità, la giusta remunerazione del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro rappresentino una condizione non derogabile. Per questo il Masaf sta innanzitutto lavorando per il rafforzamento del potere contrattuale delle imprese agricole, la distribuzione del valore lungo la filiera e l'adeguata remunerazione delle produzioni agricole, perché si riflettano direttamente sulla possibilità di offrire migliori condizioni agli occupati del settore. In questa direzione, lo scorso dicembre abbiamo potenziato la misura dei contratti di filiera con risorse pari a ulteriori 2 miliardi in sede di riprogrammazione del PNRR. L'obiettivo è quello di favorire l'integrazione tra imprese e settori produttivi per garantire la competitività, senza incidere negativamente sul contenimento dei costi di produzione, con particolare riguardo alle condizioni della manodopera. A questo si aggiunge un controllo più incisivo sulle pratiche commerciali all'interno del sistema agroalimentare, attuato tramite le azioni di contrasto alle pratiche sleali. Allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori abbiamo destinato risorse senza precedenti per la sicurezza del lavoro agricolo e per l'introduzione di innovazioni tecniche di avanguardia. L'obiettivo di questo Governo è diminuire i rischi e abbattere la piaga delle morti sul lavoro, scopo che dobbiamo raggiungere con strumenti nuovi e più potenti, poiché l'eredità che ci è stata lasciata dai Governi precedenti appare in questo senso insufficiente. Voglio ricordare che la rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS nel lontano 2014 e che oggi necessita di una profonda revisione, non è stato uno strumento evidentemente efficace. Basta guardare i numeri attuali di adesione a questo programma. Dunque, se un problema esiste riguarda non certo la volontà di questo Governo, ma l'efficacia di uno strumento disegnato male all'origine. In tal senso è opportuno ricordare il nuovo bando INAIL con uno stanziamento più che raddoppiato (da 35 più che raddoppiato (da 35 a 90 milioni di euro) per incentivi diretti all'acquisto di mezzi per l'agricoltura più sicura. Con questo strumento il Governo ha voluto promuovere e valorizzare le aziende virtuose che puntano sulla sicurezza del lavoro e sulla salute dei dipendenti. La misura del PNRR per la meccanizzazione in agricoltura contribuisce con 500 milioni di euro per ammodernare i macchinari, con lo scopo di aumentare la produttività e migliorare la sostenibilità ambientale del settore. In questo ambito, in maniera complementare opera il Fondo innovazione ISMEA, con 100 milioni di contributi a fondo perduto nel 2024, che mira a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione fino a 500.000 euro nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la diffusione di migliori tecnologie disponibili per modernizzare le imprese e renderle competitive, per avere un valore maggiore da ridistribuire in maniera equa all'interno della filiera, a cominciare ovviamente da coloro che operano all'interno dell'azienda come operai e lavoratori. Il rafforzamento della filiera, la correttezza delle pratiche commerciali, il sostegno all'innovazione rappresentano punti di riferimento per lo sviluppo di un sistema agricolo più equo, legale e competitivo, in grado di garantire l'assenza di comportamenti sleali e dello sfruttamento dei lavoratori.

prendere quei fondi, visto che nella Missione 5 erano stanziati proprio per quella che è la base della risposta che deve essere data ai lavoratori ridotti in schiavitù. Il Governo non dà risposte e vi è sempre il solito snocciolare i minimi fondi dati a destra e a manca, che alla fine non segnano alcun cambiamento radicale, alcuna situazione risolutiva di un problema contingente

L'infortunio è stato l'inizio di una vicenda che - ripeto - si chiama omicidio e che fa parte di un sistema. Non è un evento drammatico, non è una cosa eccezionale, non è una cosa imprevedibile: è un sistema organizzato di sfruttamento

che determina il fatto che ci possa essere un sistema di sfruttamento così organizzato che riguarda una comunità precisa e che nel nostro Paese ci sta da molti anni? anni? Forse dovremmo interrogarci se questo non è l'effetto dell'impossibilità di entrare nel nostro Paese e trovare un lavoro regolare, perché la Bossi-Fini lo impedisce, e perché i decreti flussi, così come sono stati costruiti, in realtà non permettono l'acquisizione delle condizioni effettive di soggiorno. Quei lavoratori, allora, allora, sono quotidianamente ricattabili e lo sono da anni e anni. Noi preferiamo - e tanta retorica preferisce - non vederli, ignorare la loro esistenza e pensare che siano sottraibili ai nostri sguardi, invece di domandare come si può rimediare a tutto questo e ricostruire una condizione innanzitutto di cittadinanza e poi anche di lavoro positivo. lavoro positivo. Noi non abbiamo alcuna intenzione di criminalizzare le imprese, men che meno genericamente, però ci sono delle cose che ci sfuggono: non c'è un mondo delle imprese che solleva il fatto che quella è concorrenza sleale e quindi si mette in prima fila per contrastare gli elementi di caporalato? Perché tacciono? I silenzi alla fine sono spesso degli elementi che favoriscono quel clima.

Seconda azione, già prevista dalla legge sul caporalato: quando definiamo i DURC, cioè quando si definiscono gli indici di congruità a cui le aziende non possono sottrarsi e non possono avere lavoratori che sono sommersi in nero e irregolari, perché risulta dai loro dati? La terza cosa da fare è sui controlli: noi abbiamo visto l'emendamento che avete proposto al decreto agricoltura, ma i controlli sono troppo pochi e bisogna fare i bandi subito. Non possiamo continuare a essere in una situazione in cui i controlli non ci sono e quindi - da un lato - le aziende sono convinte dell'impunità e - dall'altro - soprattutto i lavoratori non si sentono protetti e garantiti. Quei lavoratori, che sono spesso lavoratori stranieri, dovrebbero anche essere garantiti dal fatto che,

Camusso del suo intervento, che è stato particolarmente costruttivo nei toni. Così come sono stati particolarmente costruttivi nei toni e nei modi tutti i tavoli che abbiamo finora realizzato, in tempi non sospetti e prima del tragico evento, rispetto a quelle che devono essere le condizioni che pongano fine a un perdurante stato delle cose che mette in condizione di avere una situazione che garantisce poco i lavoratori, in particolare coloro che sono arrivati attraverso decreti flussi male organizzati in passato. La legge va oggettivamente rivista, perché datata, e perché mette in condizione di rischio, di pericolo e anche - come lei sottolineava - di ricatto i lavoratori, fino ad arrivare a quella tragica morte, che oggi in quest'Aula denunciamo con cordoglio tutti, di cui - come lei sottolineava - è responsabile un criminale, più che un imprenditore. È proprio il lavoro che il tavolo che abbiamo composto e che abbiamo riunito l'ultima volta alcuni giorni fa, insieme alla collega Calderone, tende a provare a sottolineare come esigenza: un rapporto non dicotomico tra imprese e rappresentanze del mondo del lavoro; una sinergia di sistema che ponga fine alle condizioni che tutti abbiamo da anni davanti agli occhi e che, al contrario di quanto auspichiamo, restano in una situazione in cui in troppi - e credo da tutte le parti - si sono voltati dall'altra parte. Abbiamo dato disponibilità come Ministero, anche rispetto a denunce anonime, di sostituirci ai lavoratori per perseguire chiunque sfrutti il lavoro, creando anche quelle condizioni di concorrenza sleale che minano la competitività delle imprese serie, che tutelano i loro lavoratori con adeguate norme di sicurezza,

insieme al Governo e a tutte le istituzioni di questo Stato, intervenire con una normativa adeguata e l'applicazione delle normative esistenti. Io non ho pregiudiziali anche rispetto a fattori incentivanti. Questo è stato l'esito del tavolo rispetto al controllo delle imprese di qualità. Visto che la volontarietà non ha portato da nessuna

di una produzione e di un fatturato dove non risultano adeguate retribuzioni e un adeguato numero di lavoratori. Ed è per questo che è stata composta una cabina che abbiamo implementato anche nelle ultime ore, con il contributo del nostro Ministero, che è solo per quota parte competente rispetto alle questioni di merito dei lavoratori, con l'intervento di AGEA che, grazie anche alle sue tecnologie di rilevamento ai contributi richiesti, ai terreni coltivati e alle produzioni che vengono in essere, può segnalare una discrasia rispetto al numero di occupati e alle norme di sicurezza che vengono poste in essere. Sono stati già annunciati alcuni interventi dalla presidente Meloni con l'anticipo delle assunzioni dei nuovi ispettori, perché ne servono tanti rispetto ai numeri anni. Quello che potevamo fare era cercare di riorganizzare anche il Ministero dell'agricoltura, riportando le dipendenze funzionali del CUFA in capo al Ministero dell'agricoltura, per avere un numero sufficiente anche di uomini delle Forze dell'ordine che potessero intervenire nei controlli. Erano rimasti, quando io sono arrivato al Ministero, 140 Carabinieri dell'agroalimentare e per tutto il Ministero dell'agricoltura. L'Ispettorato del controllo qualità e repressione frodi era arrivato a numeri da estinzione. Si è parlato di pioggia di assunzioni quando abbiamo spiegato che assumere persone nello Stato è un fatto positivo, perché ci mette in condizione di intervenire, risolvere i problemi e anche affrontare problemi che non possono essere rinviabili come quello che è stato citato. Da parte nostra, non c'è alcuna volontà di ribaltare delle situazioni, e - come ha fatto lei nel suo intervento - con

che ovviamente deve essere dimostrata con azioni concrete e cogenti, che possano migliorare ancor di più le condizioni in essere per arrivare a una Nazione che si possa fregiare magari di un *record* positivo, in cui non ci siano più morti sul lavoro ed episodi di questa natura. Ho apprezzato quello che lei ha detto e sottolineo ancora una volta che c'è non una criminalizzazione delle imprese, ma la volontà di stanare i criminali in ogni ambito si annidino, che si macchiano di responsabilità gravissime come quella del potenziale omicidio a cui lei ha fatto riferimento.

Non basta qualche impegno - lo apprezziamo, ma è troppo generico - per combattere il mostro del caporalato. Stiamo parlando di una condizione in cui i lavoratori e le lavoratrici sono ridotti in schiavitù: sfruttati, sottopagati, costretti a vivere in alloggi fatiscenti, minacciati e anche ammazzati. Oggi dite che assumerete nuovi ispettori, ma sono mesi che presentiamo emendamenti perché si assumano.

speriamo che abbiate almeno la lungimiranza di accettare, nella discussione sui vostri emendamenti, le proposte che i colleghi della Commissione agricoltura presenteranno perché il numero sia adeguato. Parliamo comunque di assunzioni che lei sa bene, avendo fatto anche scadere le graduatorie, saranno tra tempi non brevissimi. non basta, signor Ministro. Bisogna fare molto di più come, ad esempio, creare condizioni di vantaggio per le imprese che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità: sono pochissime quelle che hanno aderito, perché gli incentivi non sono adeguati e perché la stessa cultura sta diventando complicata per quanto riguarda la legalità e la qualità del lavoro. Iniziamo ad esempio a dire, signor Ministro, che informiamo immediatamente adeguatamente tutti i consumatori

Iniziamo anche dire che le imprese che non aderiscono, perché non sono in regola per poterlo fare, non partecipano più, ad esempio, a alcun appalto pubblico.

Penso a Latina: di quei 200 milioni non spesi, oltre quattro dovevano andare a Latina, per creare condizioni anche di vita, di abitabilità, degne di essere umani. Che fine hanno fatto, signor Ministro? Non se ne ha traccia, è tutto bloccato e quei lavoratori continuano a vivere in condizioni disperate. Vada a vederli. Vada a Latina, vada a Foggia e veda anche le fogne a cielo aperto. Sembra un altro Paese, non certo il nostro. Allora, signor Ministro, se vogliamo davvero affrontare la tragedia del caporalato, bisogna farlo con strumenti, risorse, con serietà, a partire dal superamento della legge

ogni dieci lavoratori immigrati che arrivano col *click day,* forse solo due, nella migliore delle ipotesi, sono regolarizzati? Questi dati non li abbiamo solo noi, ma li ha anche lei, signor Ministro. E poi bisogna metterci testa, cuore e risorse, perché è una battaglia di civiltà da vincere in questo Paese e noi faremo di tutto perché questo avvenga. Sabato e martedì abbiamo partecipato a due grandi iniziative insieme ai lavoratori immigrati, insieme alla comunità indiana. Ascolti quelle parole, signor Ministro, e finalmente promuova lei, all'interno del Governo, anche presso gli altri Ministeri coinvolti, azioni vere, affinché quello che è successo non si ripeta più.

*(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, gli ultimi eventi climatici, con l'alternanza di precipitazioni, brevi o intense, siccità e alluvioni consegnano l'immagine di un Paese letteralmente diviso a metà, contemporaneamente colpito da gelate e alluvioni al Nord e da grave siccità al Sud. La situazione è di assoluta emergenza a livello nazionale. L'ondata di maltempo che ha investito soprattutto il Nord del Paese ha comportato l'allagamento dei terreni agricoli, rendendo impossibili le semine interferendo nel processo di maturazione delle coltivazioni primaverili ed estive, mentre al Sud la siccità sta mettendo in seria difficoltà il comparto cerealicolo e ortofrutticolo. Lo scenario rappresentato è la riprova della tropicalizzazione del nostro clima, con un aumento costante delle temperature e sfasamenti stagionali con brevi ed estremamente intense precipitazioni. Siccità, alluvioni, cuneo salino, sono tutti fenomeni interconnessi che si stanno acutizzando e influenzando a vicenda, minando il settore primario al punto da renderlo il più esposto e il più debole. Negli invasi di Puglia, Basilicata e Sicilia, la situazione mostra valori di riempimento più bassi rispetto al volume utile di regolazione, mentre al Nord abbiamo avuto un aumento di precipitazioni, precipitazioni, arrivando a un *surplus* del 42 per cento rispetto al periodo 2011-2022. Le imprese agricole sono in prima linea nel vedere e misurare sul campo gli effetti dei cambiamenti climatici: sono le sentinelle in grado di captare i primi segnali e i danni prodotti sono esse stesse, al contempo, in difficoltà e noi abbiamo il compito oggi di aiutarle. Le Regioni più colpite al Nord sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia. Segnalo ad oggi - sono dati che ho avuto questa mattina - che in Piemonte le prime stime sui danni subìti in questo periodo superano i 215 milioni di euro, a partire dai cereali a paglia, in quanto avranno destinazione diversa da quella alimentare. (due terzi della produzione di ciliegie è stata persa), quello vitivinicolo e quello zootecnico per mancanza di fienagione e soprattutto quello risicolo per mancanza di semine. Il tema è quello delle polizze assicurative, e lei lo sa bene. C'è difficoltà anche sui fondi mutualistici. Occorre anche adottare opportuni interventi per incoraggiare la crescita del sistema assicurativo nel nostro Paese Chiediamo semplicemente, signor Ministro, se può promuovere un'iniziativa

dell'implementazione assicurativa. Ringrazio il collega Bergesio e il Gruppo Lega per aver sollevato un importante quesito che offre l'opportunità di aggiornare l'Assemblea sulle misure adottate dal Governo Meloni per contrastare le ripercussioni degli eventi siccitosi e sul resto delle crisi che riguardano i nostri agricoltori. Poiché la deliberazione dello stato di emergenza nazionale relativo ad eventi siccitosi è competenza strettamente posta in capo al Ministero per la Protezione civile e per le politiche del mare, poiché il coordinamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali per la risorsa idrica sono di competenza poste in capo al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, risponderò mi scuserete - per quanto di mia competenza, ovviamente sapendo che i colleghi di Governo sono più attivi di me, certamente, rispetto a queste priorità e io comunque resto nella disponibilità di offrire qualsiasi contributo attivo. Con uno dei primi decreti-legge adottati nel 2023, il Governo Meloni ha infatti istituito una cabina di regia dedicata alla gestione della crisi idrica, coordinata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole senatore Matteo Salvini, che ha provveduto alla nomina del dottor Nicola Dell'Acqua come commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti contro la scarsità idrica. Queste due azioni hanno congiuntamente permesso di avere una visione coordinata e integrata degli interventi necessari. Nella legge di bilancio del 2024 abbiamo provveduto a istituire un fondo emergenza in agricoltura, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, finalizzato a sostenere le imprese agricole e della pesca colpite da eventi non prevedibili. Attraverso specifici decreti del nostro Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno presto definiti i criteri di accesso al fondo, individuando i riferimenti delle condizioni di crisi, i beneficiari e la modalità di erogazione delle risorse, al fine di offrire un supporto concreto alle imprese interessate il prima possibile, ovviamente anche con il coinvolgimento della rappresentanza delle Regioni, per comprendere, rispetto alle risorse date, quali il sistema agricolo ritiene maggiormente importanti come esigenze. Meritevole di menzione è anche il decreto agricoltura, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 maggio scorso ed ora in corso di conversione proprio qui in Senato, con il quale abbiamo ulteriormente rafforzato i poteri del commissario dell'acqua, per garantire l'implementazione delle misure più urgenti, strutturali e gestionali, per contrastare la scarsità di acqua, ma soprattutto per intervenire in termini strategici a compensare quello che non è stato fatto negli ultimi perché di questo parliamo. Sempre nel medesimo provvedimento abbiamo inoltre destinato 102 milioni di euro alla realizzazione degli invasi e al risparmio idrico negli usi agricoli e civili; risorse che provengono dalla rimodulazione del piano straordinario per il settore idrico. Il quadro delle risorse previste è inoltre destinato ad essere implementato di altri 15 milioni per la sola Regione Siciliana, in virtù dell'entità del tutto particolare della crisi dovuta alla siccità di quest'anno. La gravità della situazione in Sicilia richiede un intervento specifico. In collaborazione con il Governo della Regione Siciliana, abbiamo attivato un sistema di raccordo costante per assicurare che le risorse approvate, approvate, anche all'atto della conversione del decreto agricoltura, entrino immediatamente nella disponibilità degli agricoltori. Il Governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per dodici mesi, in relazione al *deficit* idrico della Regione Siciliana, stanziando 20 milioni di euro per sostenere i primi interventi sul territorio. A margine di questi interventi, ricordo la massima disponibilità del Ministero nella valutazione e approvazione delle richieste di declaratoria di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale a cui lei faceva riferimento - e che devono necessariamente pervenire però al Governo su indicazione delle Regioni. Queste iniziative fanno parte dell'impegno che, come Governo Meloni, stiamo mettendo in campo per tutelare gli agricoltori italiani su ogni fronte; un impegno che non si esaurisce nel rispondere a quella che viene definita un'emergenza, ma che continua dando risposte di lungo periodo per affrontare questi problemi ormai endemici. Le casse dello Stato permettono pochi interventi rispetto a quanto ne avremmo necessità. Per questo abbiamo coinvolto il settore bancario con il protocollo d'intesa con il gruppo Intesa, ma altri ne seguiranno con il sistema bancario. Sono stati messi per il triennio 20 miliardi a disposizione del sistema agricolo e dell'agroindustria, con un sostegno per riuscire ad attivarli senza

tassi e per intervenire con la moratoria, che coinvolgono anche il sistema bancario. Mai nulla è sufficiente in sostegno dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, dei nostri pescatori, perché per noi, per questo Governo, sicuramente una priorità sulla quale insieme continueremo ad intervenire in maniera decisa, sperando che gli errori del passato, anche in termini economici, non ci mettano in condizione di rallentare troppo quello che dovrà essere lo sviluppo, in Italia e in Europa, di un nuovo concetto di centralità del nostro mondo produttivo e delle imprese, perché significa lavoro e ricchezza per il popolo italiano.

importante. È la cura dei dettagli che alla fine fa i grandi risultati in tutti i settori. Io credo che questo settore così importante del nostro Paese abbia oggi la possibilità di fare un salto di qualità. Conosciamo bene le norme che sono contenute nel decreto-legge che in questo periodo è all'attenzione della nostra Commissione. Sul tema delle assicurazioni in agricoltura, però, sono fondamentali i ristori e dare il giusto margine di valore a quello che hanno gli agricoltori. È stato fatto un passo notevole in avanti con Agricat. Il Fondo di solidarietà nazionale si è aperto anche in momenti particolari. Apprendo - e mi fa veramente piacere - che si è attivato il percorso dello stato di calamità e di emergenza per la Regione Lombardia e anche per la Regione Sicilia. Credo che questa sia una grande opportunità per tutti. Ho visto che in questi giorni sono emersi i dati relativamente alla cabina di regia della crisi idrica. Gli investimenti di 950 milioni sono messi all'attenzione dei nostri operatori, dei consorzi di tutti gli agricoltori a livello nazionale dell'idropotabile: anche questa è una risposta importante che coinvolge molti Ministeri. Dall'altra parte, c'è il piano strategico che, per la prima volta nel nostro Paese, contempla richieste per oltre 13 miliardi di euro,

produttori e la ricerca. Come non stigmatizzare poi ciò che è avvenuto solo pochi giorni fa a Pavia? Un campo dove c'era il primo esperimento a terra delle tecniche di evoluzione assistita è stato massacrato da

quasi all'unanimità. È stato un atto assolutamente antidemocratico, a dimostrazione di come ci siano ancora sacche che credono che l'agricoltura debba essere qualcosa più vicino alla sindrome di Heidi che alla vera modernità. Su questa discussione oggi si si inserisce anche il G7, che lei ha giustamente annunciato e ha voluto fortemente fare in Sicilia, terra meravigliosa, nell'isola di Ortigia, dove proprio la prima settimana di settembre si continuerà a discutere del futuro, anche mondiale, dell'agricoltura, di quale visione dare all'agricoltura. Si farà mettendo assieme per la prima volta pesca e agricoltura; si dibatterà se se l'agricoltore sia o meno un bioregolatore (quello che noi diciamo da sempre); se la tutela della pesca e dei pescatori sia centrale per le politiche agricole europee, ma anche mondiali; se ci si debba concentrare più sulla produttività, per dare in fondo risposta anche a un mondo che cresce in termini demografici e capire come faremo a dare da mangiare di più e meglio a tutti i prossimi cittadini. Soprattutto, si dibatterà su quelli che sono stati i nostri cavalli di battaglia, per esempio il no deciso al cibo sintetico, il sì alle tecniche di evoluzione assistita *(Applausi)*, che ci hanno posti all'avanguardia nel mondo. Qualcuno ci diceva che o prima il Presidente della Repubblica non l'avrebbe firmata o poi in Europa ce l'avrebbero cassata. In realtà, tanti sono quelli che oggi seguono l'indirizzo dell'Italia, grazie anche un nuovo approccio verso l'Europa che abbiamo avuto. Signor Ministro, noi le chiediamo di delineare quali sono i contenuti che l'Italia porterà e quali sono i risultati che lei si attende da un

foreste*. Signor Presidente, mi scusi anche dalla lunghezza degli interventi, ma siamo contenti che sia tornata così centrale la discussione dell'agricoltura nel nostro Parlamento da quando c'è questo Governo. Desidero ringraziare il senatore De Carlo e tutto il Gruppo Fratelli d'Italia per la sottolineatura delle politiche del Governo, che ovviamente da uno dei partiti di maggioranza viene condivisa. Si auspica, anzi, di poter dare ancora più corpo alle programmazioni che vedono, ancorandoci a valori profondi che fanno parte della nostra cultura alimentare, valorizzare le innovazioni tecnologiche, (TEA). Oggi voglio esprimere la mia solidarietà rispetto all'attentato di ecoterroristi al campo sperimentale, autorizzato dall'Europa, che ci avrebbe permesso di rispondere anche alle questioni legate al riso, che cercheremo però anche in questo decreto di garantire nella sua prosecuzione, perché l'Italia non si ferma rispetto a chi compie atti di quella natura. Allo stesso tempo occorre contrastare quelle derive che vorrebbero trasformare il nostro modello di produzione alimentare, che è anche garante dell'ambiente e del territorio, in qualcosa di diverso. Qualcuno ha immaginato che potessimo potessimo avere un futuro in cui i terreni agricoli potessero ospitare pannelli che impediscono la produzione per finanziare energia dei laboratori che producono cibo. Non è il mondo a cui noi ci arrenderemo e su questo proprio nel G7 ci sono state parole importanti, già a Savelletri, a Brindisi,

dell'Africa, particolarmente giovane, che deve essere sostenuta ed aiutata per uno sviluppo che garantisca autosufficienza alimentare, ma anche ricchezza attraverso la valorizzazione dei loro prodotti, sulla base di tecnologie e formazione che i Paesi più sviluppati e democratici devono offrire, in una *partnership* che non sia né caritatevole, né predatoria, come in passato è avvenuto, ma che permetta, come Mattei fece, di trattare l'Africa in pari condizioni rispetto a come l'Europa tratta le altre Nazioni del suo consesso. Sono contento che lei abbia sottolineato il risultato straordinario del G7 pugliese, al quale hanno partecipato il sommo Pontefice e Modi, il Presidente della Stato più popoloso del pianeta, che ha avuto una rilevanza di carattere internazionale e oltre ogni aspettativa, valorizzando il nostro territorio e le nostre produzioni. Ce ne sarà un altro, ovviamente di tono inferiore in termini di verticalità di partecipazione (è insuperabile quello organizzato dalla presidente Meloni), ma di compensare con il periodo più lungo di permanenza sull'isola di Ortigia. Abbiamo scelto Siracusa: luogo della tradizione, luogo della scoperta della cultura per la nostra Italia, grazie ai greci in origine. Questo ci permetterà di garantire una discussione che proseguirà e

giovani, anche grazie ai nostri ragazzi che possono, con le loro competenze fornite da scuole eccezionali come gli istituti agrari, dotare i ragazzi africani, perché possano scegliere anche se rimanere nelle loro terre, vicino alle loro famiglie, piuttosto che essere costretti ad emigrare per fame. Abbiamo però voluto affiancare al G7, la cui durata è di tre giorni, altri giorni: dal 21 al 29 settembre a Ortigia avremo la più grande esposizione del sistema agricolo e agroalimentare che in Italia si sia svolta probabilmente negli ultimi decenni, per la centralità di quella Regione; vedrà la partecipazione delle Regioni, delle grandi imprese, della grande qualità italiana, e potrà essere la vetrina del nostro sistema che auspica essere la guida per una politica di sicurezza alimentare che non si risolva con cibo per tutti, ma con buon cibo per tutti, al di là della ricchezza e del censo di chi si potrebbe permettere sempre un'alimentazione ottimale, condannando condannando magari gli altri a mangiare cose che noi riteniamo invece disprezzabili e che riteniamo non debbano essere considerate cibo, ma eventualmente carburante per andare avanti.

non vediamo l'ora di iniziare questo G7, per cui abbiamo accorciato i tempi. In realtà sarà verso la fine di settembre, ma sarà uno degli strumenti che questo Governo continua a mettere in campo per spiegare sua filosofia. Spesso, quando si parla di politica, ci si interroga e ci si chiede se esiste o meno una visione. A volte la visione è contundente e talvolta si pensa solo a quello che dovremmo fare oggi o domani, e dietro lo slogan magari c'è poco o nulla. In realtà la visione di questo Governo, di questa maggioranza e di questo Gruppo, soprattutto in agricoltura, viene dal retaggio della precedente legislatura ed è quella di un'agricoltura fatta per produrre di più e meglio, per garantire cibo di qualità a tutti, per far sentire gli agricoltori parte di un sistema straordinariamente fondamentale per l'Italia, di quel *made in Italy* che oggi tutto il mondo ci copia, di quel sistema che consente aziende a valore aggiunto straordinario, quel sistema che oggi è messo sempre fortemente in difficoltà, una volta dalla crisi mondiale, una volta dalla crisi energetica, un'altra volta dalla crisi climatica. Anche su questo abbiamo dato in Commissione risposte dirette, attuando per esempio, con il collega Bergesio e con gli altri colleghi della Commissione, un'indagine conoscitiva per capire se abbiamo gli strumenti per monitorare ciò che accade.

scorsi, negli ultimi vent'anni, abbiamo pensato che l'agricoltura fosse meglio non farla, che gli agricoltori dovessero fare i giardinieri e che noi dovessimo acquistare i prodotti e le materie prime da altre parti del mondo dove costavano meno e quindi non ci siamo dotati degli strumenti per capire se eravamo moderni o no e non sapevamo come affrontare le crisi. Oggi, invece, abbiamo consapevolezza dell'importanza e della centralità dell'agricoltura, per cui tutto ciò che faremo è funzionale a riuscire a sostenere i nostri agricoltori per produrre di più e produrre meglio, con tanta innovazione, perché lo dico sempre: la nostra forza sono le tradizioni, ma le nostre tradizioni sono innovazioni che ce l'hanno fatta.

Signor Presidente, gentile ministro Bernini, come lei ben sa, la ricerca scientifica e tecnologica costituisce un volano per la crescita economica e sociale del nostro Paese ed è pertanto necessario rendere maggiormente competitivo il sistema della ricerca italiano sulla scena mondiale, con interventi mirati che garantiscano sia l'attrattività che la sicurezza. Le opportunità di formazione e di crescita personale offerte in altre parti del mondo inducono alcuni giovani studiosi italiani a scegliere di ampliare all'estero il proprio bagaglio di competenze. Questo è un fatto positivo, se poi almeno una parte di loro mette a disposizione la propria crescita professionale degli istituti di ricerca e delle università italiane. Occorre quindi che le istituzioni promuovano l'innovazione in ogni ambito, attraendo ricercatori dall'estero e trattenendo i migliori talenti all'interno del nostro Paese, arginando e contrastando quella che viene definita fuga dei cervelli. Nondimeno i dati ci confermano che il settore pubblico in Italia guida e stimola ancora gli investimenti in ricerca e sviluppo, a differenza di quanto avviene in altri Paesi industrializzati, dove l'innovazione è trainata dal privato. Per questo è essenziale incentivare la creazione di infrastrutture avanzate e investire sulle tecnologie emergenti. Così come è importante individuare i modi più opportuni per facilitare il trasferimento tecnologico della ricerca pubblica al mondo delle imprese, come sta facendo proprio il PNRR di sua competenza. Sappiamo che lei, gentile Ministro, sta lavorando molto seriamente e con generosa competenza in questa direzione, per cui le chiediamo quali misure abbia adottato o intenda adottare per rendere sempre più sicuro e competitivo il sistema della ricerca, per far fronte alle sfide globali che vedono l'Italia interfacciarsi con gli altri *partner* europei e internazionali nel campo dell'innovazione, delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale.

enorme, però cercherò di sintetizzare quello che abbiamo fatto sino ad ora come Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (perché ci occupiamo anche di accademie, conservatori e scuole di *design*), rispetto ad una aspettativa giustamente altissima da parte dei soggetti che si rivolgono a noi. Noi siamo una fabbrica che produce futuro, siamo un *hub* che produce costantemente futuro; siamo i depositari di aspettative, talenti, sogni di studentesse e studenti. Come fare, cosa mettere in atto? Prima di tutto, nelle interrogazioni che mi hanno preceduto usare il cuore (quindi di saper intercettare i talenti), la testa, di valutare la qualità, la flessibilità e l'attualità dell'offerta formativa, ma soprattutto di prevedere finanziamenti.

tema di smentita. Tutto ciò riguarda l'*housing*, cioè gli studentati, perché i capaci e i meritevoli devono non solo poter studiare in un'università, ma anche avere un luogo dove poter dormire e studiare fisicamente.

attraverso le quali si fanno rimanere o tornare i ricercatori che se ne sono andati, magari accompagnati anche da ricercatori stranieri che vengono a fare attività di ricerca da noi. Su questo, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo investito 11 miliardi.

e tecnologie quantistiche, recupero della biodiversità, tecnologie come la mobilità sostenibile, terapie geniche e farmaci a tecnologia a RNA,

droni, satelliti, genomica, metabolomica. Noi su questo stiamo investendo con un centro nazionale *agritech,* che ha come capofila l'Università Federico II di Napoli. È in questo modo che noi faremo tornare i nostri cervelli, accompagnati da altri cervelli cervelli stranieri che devono venire a studiare, a lavorare, a vivere e a consumare in Italia. Intendo consumare cultura, perché noi siamo il luogo dove tutto è nato. Organizzeremo a Bologna

cioè di come le infrastrutture strategiche e gli investimenti che stiamo facendo ora (infrastrutture e investimenti che significano futuro per le nuove generazioni, non spesa corrente) possano non solamente essere un'occasione, un modo per studiare, un riflesso immediato sull'impresa, perché tutta la ricerca di base ha un'applicazione sull'impresa e un'applicazione che può migliorare la qualità della vita di tutti noi e aumentare la qualità dei nostri anni; insomma farci vivere di più e meglio. Senatore, lei ha un orologio che è proprio il frutto di una ricerca che magari è partita in un laboratorio di astrofisica ed è finita nel suo telefonino, nei suoi *microchip*, nelle sue nanotecnologie, che rappresentano un modo per vivere di più e meglio e avere una qualità di vita migliore. Questo è il nostro obiettivo, come Ministero dell'università e come Governo. Questi sono, naturalmente, i traguardi che abbiamo raggiunto ad oggi. Grazie, ministro Come imprenditore di un settore che ha un *business* di tipo tradizionale, ho visto come l'innovazione in azienda giochi un ruolo fondamentale per far crescere sia la dimensione che l'*export*. È un tema di interesse generale che riguarda il vasto tessuto di piccole e medie imprese italiane che usufruiscono di quell'interazione pubblico-privato nei progressi tecnologici. Questo significa per le nostre aziende diventare più competitive con il resto del mondo. Ecco perché mi sento di ringraziarla per la risposta, che ha centrato il tema, e per il lavoro importante che avrà al G7 scienza e tecnologia di luglio in Emilia-Romagna, dove lei guiderà il tavolo dei grandi della Terra su questo tema. Incentivare la ricerca, sia pubblica che privata, serve a creare un ambiente dove crescono i talenti, prospera l'impresa e migliorano le opportunità per tutti i cittadini.

Signor Presidente, volevo ricordare con pochissime parole Stefano Navarrini, illustratore, grafico, artista scomparso in queste ore e che tanto ha dato all'editoria italiana (a giornali come «la Repubblica», «il Messaggero», «la Stampa», «Europa») che è stata la sua famiglia disfunzionale e cara come tutte le famiglie. Stefano sembrava un fumetto uscito dalla sua penna essenziale, elegante, stralunata; un uccello che nessuna stanza di giornale riusciva a tenere prigioniero. Uomo mite dalle improbabili imprecazioni, di un altro mondo, di un'altra musica che non questa di convenienza e banalità. Mancheranno la sua invenzione del possibile, i suoi pomeriggi in stanza con Giulio e Cinzia, le visite timide di Antonella, la sua grafica internazionale. Il «New Yorker» non sa che si è perso. *(Applausi)*.